il metodo infatti, ancora una volta, il Senato è chiamato ad approvare in maniera frettolosa un altro di quei provvedimenti contenitore cui siamo abituati da parecchi mesi. Tante sono le materie contenute in questo provvedimento; basta leggere il nome del disegno di legge (sviluppo economico, semplificazione, competitività e riforma del processo civile) per capire che ci troviamo di fronte ad un altro di quei calderoni di norme che, a volte, rischiano di disorientare il Parlamento, pregiudicando la qualità del confronto parlamentare e delle proposte e portando le Camere ad approvare atti quasi al buio, senza avere tempi ragionevoli per lo studio delle norme in esso contenute. Il tema che sembra emergere come centrale da questo pentolone di norme è, ovviamente, la riforma del processo civile; un tema di grandissima rilevanza ed urgenza per il nostro Paese - come più volte abbiamo dal cui destino dipende non solo la funzionalità della macchina giudiziaria, ma anche la garanzia di un sistema economico e sociale efficiente. In questo ambito noi rivendichiamo il ruolo di mediazione che abbiamo tentato di svolgere sul campo in materia della giustizia, in particolar modo di quella civile, formulando alcune proposte concrete, facendoci promotori di iniziative e di documenti e cercando di dare un contributo costruttivo nelle Aule parlamentari, nei limiti in cui ciò ci è stato consentito, atteso il metodo seguito nell'esame e nell'approvazione di determinati provvedimenti. Proprio per questi motivi e perché abbiamo a cuore, ritenendola indifferibile, una riforma mirata del processo civile come degli altri riti, avremmo voluto affrontare questo argomento con maggiore tempo a disposizione

provvedimenti. Proprio per questi motivi e perché abbiamo a cuore, ritenendola indifferibile, una riforma mirata del processo civile come degli altri riti, avremmo voluto affrontare questo argomento con maggiore tempo a disposizione e con dinamiche parlamentari che ci avessero permesso di comprendere meglio il contenuto dei testi che ci vengono presentati. di fronte a questo modo di procedere e ad una pratica che è diventata ormai una costante di questo Governo, il merito non può che finire in secondo piano rispetto al metodo. Indicativo delle forzature cui sempre più spesso quest'Aula va incontro è il fatto che si sia pensato di rendere questo scatolone *omnibus* di norme anche un collegato alla finanziaria, per inserirci tutto ciò che mancava in una manovra lo ricordo - è stata varata prima della crisi finanziaria e quindi, sostanzialmente, è divenuta archeologia fiscale già diversi mesi fa. Al suo interno, oltre ad una parte di riforma del processo civile, sono contenuti interventi sui Vigili fuoco, sui rifiuti, sui precari, sui dirigenti pubblici, sui Comuni e su tanto altro ancora.

sui precari, sui dirigenti pubblici, sui Comuni, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un grande calderone che rientra in una strategia mirata di confusione, magari volta a infilare a tranello qualche emendamento. In più, ci siamo trovati nel paradosso di dover affrontare il tema della giustizia civile senza che il testo potesse essere esaminato diffusamente dalla Commissione giustizia, ridotta a semplice erogatrice di un parere consultivo a Commissioni che non si sono mai occupate - e non si possono occupare - di questo argomento, ovvero di un tema estremamente delicato e importante per la giustizia italiana, quale quello della riforma del processo civile. Ciò detto, noi riteniamo giusto e condivisibile il principio di velocizzare il lavoro parlamentare, ma ci sono dei limiti che ovviamente tale velocizzazione deve incontrare quando l'esigenza di dare tempi certi sull'approvazione dei provvedimenti si scontra con la necessità di rendere rendere qualificati questi provvedimenti. Prendiamo atto che il Governo, per sua stessa ammissione, non ha pensato di procedere a una totale rivisitazione del processo civile. di per sé un elemento negativo se si pensa ad alcuni aggiustamenti mirati ed efficaci: non credendo che ci siano le condizioni per fare riforme epocali, si può comunque cercare di fare dei passi avanti. Quindi, prendiamo atto della necessità di intervenire su questa materia e a tal fine abbiamo cercato di dare - nei limiti in cui ci è stato consentito - il nostro contributo, certo registrando la difficoltà che si possa affrontare un tema con la tecnica di tagliare e pezzi provvedimenti importanti per il Paese, inserendoli di volta in volta in atti parlamentari diversi, in maniera parziale, senza guardare al contesto generale e senza a consentire un adeguato confronto di merito in Parlamento. Uno dei temi più controversi del disegno di legge è certamente quello che riguarda il filtro in Cassazione, la previsione di un giudizio di ammissibilità del ricorso. Si tratta di una circostanza sulla quale abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra contrarietà per la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, per la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, posto che, com'è noto, nel prevedere la proponibilità del ricorso per Cassazione avverso avverso tutti i provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 111 non contiene alcun limite, con la conseguenza che l'inserimento di un vaglio preliminare di ammissibilità, ovvero di inammissibilità, sembra in contrasto non solo con i principi contenuti nella norma costituzionale che riguardano il giusto processo, ma con il principio più generale della garanzia del diritto di difesa, di cui all'articolo 24. Peraltro, la Corte costituzionale sembra orientata nel senso della illegittimità di norme che prevedano filtri di ammissibilità. Quindi, l'articolo 360-*bis*, proposto dalle Commissioni, dal nostro punto di vista sconvolge il sistema costituzionale fissato dalle norme che abbiamo richiamato. Abbiamo presentato una serie di proposte per un processo civile equo e funzionale, convinti che per rifondare la giustizia nel nostro Paese occorra ripartire da princìpi e criteri chiari: giudizi più rapidi, razionalizzazione delle risorse, semplificazione e ragionevolezza del sistema, perché spesso la lentezza dei processi e l'incertezza con cui vengono portati avanti finiscono per compromettere la ragionevolezza stessa del processo. in particolare in un settore come il civile, significa eliminare le lungaggini formali e la pluralità dei riti che contribuiscono a rendere interminabile un processo. Condividiamo, quindi, la necessità di ridurre e semplificare procedimenti civili e riteniamo che la filosofia che aveva condotto via via ad aggiungere regole a regole, quasi in una sorta di superfetazione normativa, quella cioè secondo cui per avere decisioni più rapide una delle strade da percorrere fosse quella di modulare il rito sul tipo di controversie, sia una filosofia che vada superata. E nel testo - ne dobbiamo dare atto anche alla maggioranza - vi sono evidenti tracce della esigenza di superare questo modo di affrontare le controversie. Siamo, viceversa, fortemente perplessi sulla introduzione della testimonianza scritta che, certo, non rientra nella cultura giuridico-processuale italiana. In ogni caso, la sua introduzione presuppone un sistema ed un ordinamento dell'avvocatura che ancora oggi non esiste in Italia. Infine, va ricordato che l'analoga previsione introdotta dall'articolo 116-*ter* del codice di procedura civile per l'arbitrato ha suscitato e promosso un dibattito critico estremamente ampio. Fra le proposte che abbiamo fatto in questa materia, che non ci è stato dato modo e possibilità di affrontare per le strettoie del dibattito parlamentare, vi è quella dell'introduzione del giudice monocratico per tutto il primo grado del giudizio civile, al contempo alle esigenze della riduzione dei tempi e della riduzione delle risorse necessarie. Del resto, se oggi nel nostro Paese un unico magistrato può decidere l'arresto di un cittadino, non capiamo come non possa essere in grado di decidere su un divorzio o su un fallimento.

È poi praticamente impossibile esprimere un giudizio su tutti i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge. Confermiamo le nostre perplessità per l'incremento delle competenze del giudice di pace, che se da una parte libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, dall'altra inflaziona la domanda giudiziale e sobbarca ancor più di lavoro figure fondamentali del nostro ordinamento alle quali, comunque, non si stanno corrispondendo adeguate tutele e riconoscimenti. Anche stavolta immancabile costante immancabile costante di ogni provvedimento del Governo - e quindi anche di questo - è l'utilizzazione a piene mani dei fondi FAS. Questa volta serviranno al Governo per garantire la banda larga nelle aree sottoutilizzate. Ci chiediamo, e soprattutto vi chiediamo se, in zone in cui mancano servizi essenziali e le infrastrutture sia serio e ragionevole dare precedenza alla banda larga piuttosto che ad altre ben più importanti priorità. Non è la prima volta che ciò accade. Vi sono state promesse in tal senso: tutte fino ad oggi puntualmente disattese. Nonostante i molti elementi negativi presenti nel testo, noi riteniamo che sia necessario astenersi. Una decisione che nasce dalla consapevolezza che una riforma del processo civile - che è l'elemento prevalente di questo disegno di legge - sia imprescindibile e indifferibile nel nostro Paese e che quel poco che è stato fatto possa comunque rappresentare un punto di partenza per un cambiamento lungamente atteso dai cittadini, sulla cui attuazione non ci possono essere dubbi né ripensamenti. La nostra, quindi, è una scelta in linea con l'atteggiamento fino ad oggi tenuto, che tenta di privilegiare il confronto di merito, ovviamente nei limiti in cui ciò è possibile. Un atteggiamento che tiene anche conto della perdurante crisi economica, resa in tutta la sua drammaticità dai recenti dati ISTAT - che vedono il nostro PIL perdere un punto percentuale nel 2008 - e dalle stime degli economisti, che per il 2009 prevedono una contrazione ancora più evidente del prodotto interno lordo. Un Paese che va indietro invece di andare avanti è un problema per tutti, senza distinzioni di partiti. Per questo non ci mettiamo di traverso con un voto contrario, ma non potete chiederci di votare a favore di un provvedimento il cui *iter* è stato portato avanti in questa maniera. State riducendo la nostra attività parlamentare a quella di semplici passacarte. Questo modo di legiferare creerà dei problemi molto seri, perché alla fine non si avrà una visione generale della tenuta del nostro ordinamento e non avremo la coerenza del sistema normativo, che in un Paese civile e serio è necessaria soprattutto quando si vogliono fare riforme fondamentali.

così come avevo annunciato in sede di discussione generale, il nostro voto sarà contrario.

per arrivare a conclusioni condivise, sulle quali peraltro già in passato vi era stata condivisione. Sappiamo benissimo, ed è giusto il richiamo che ha fatto il senatore D'Alia, che

proponendo al Senato di riprendere il lavoro che si era purtroppo interrotto una volta giunto alla fase conclusiva.

Con l'articolo 26‑*quater*, di cui ieri si è discusso dopo il parere richiesto alla 5a Commissione, si è introdotta la delega per la riforma del processo amministrativo, materia complessa che necessitava di una particolare attenzione,

Invece, con questo provvedimento si prevede, in maniera che riteniamo non corretta,

interviene? Sappiamo che la legge che regola il funzionamento del Consiglio di Stato attribuisce a tale organo anche la possibilità, su incarico del Governo, di formulare testi normativi.

Così si modifica il potere che ha il Consiglio di Stato inserendo la figura degli esterni nell'elaborazione delle leggi che noi deleghiamo al Governo. Questo modifica la struttura del Consiglio di Stato, così come codificata dalla legge attuale. L'articolo 14 della legge sul Consiglio di Stato recita: «Formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo».

la compilazione». Il Ministro e il Presidente del Consiglio possono chiedere che l'affare venga discusso non da una sezione, ma in adunanza generale. Ma non si può prevedere l'inserimento di esterni nella commissione speciale, modificando nella sostanza una legge che regola il funzionamento del Consiglio di Stato! Conosciamo tutto

di tutto il Parlamento e l'articolo 111 costituzionalizzò tre princìpi: giudice terzo e imparziale, ragionevole durata del processo, garanzia del contraddittorio. Questi sono i tre princìpi costituzionalizzati nell'articolo 111, così come modificato. invece si interviene in maniera pesante con la norma cosiddetta del filtro in Cassazione, in cui sparisce uno dei princìpi costituzionali contenuto all'articolo 111, ossia il contraddittorio, di una battaglia che si è fatta per arrivare all'affermazione di un principio: la difesa e il contraddittorio devono essere garantiti con riguardo ad ogni pronuncia giurisdizionale. Invece, per quanto riguarda la fase conclusiva di un procedimento, ossia il ricorso in Cassazione, viene modificata la regola con l'esclusione del contraddittorio, per cui un organo nuovo composto da tre giudici (sappiamo che la Corte di cassazione si pronunzia con un collegio composto da cinque magistrati) può decidere composto da cinque magistrati) può decidere l'inammissibilità di un ricorso senza che la parte ne sia a conoscenza. Esiste un analogo istituto per quanto riguarda i processi in Cassazione in materia penale, ma anche in quel caso il contraddittorio viene assicurato, perché l'inammissibilità è assegnata ad una sezione - nel nostro caso la settima della Cassazione decide e delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ma alle parti viene data la possibilità di presenziare attraverso scritti difensivi; vengono avvisate le parti che il loro ricorso può essere dichiarato inammissibile e la parte può interloquire. Invece, nel processo civile si ritiene che questa stessa procedura non debba comprendere la presenza delle parti. Questa è una violazione del principio del contraddittorio sancito dall'articolo

lavoro, il processo sommario di cognizione, il processo di cognizione ordinario, il processo per il giudice di pace, il processo di appello, il rito per le procedure concorsuali, il rito per il ricorso in materia di famiglia e di minori, il rito in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rito in materia di proprietà industriale, il rito in materia di codice del consumo, tutte le procedure e i riti in materia esecutiva mobiliare e immobiliare. Ma quale semplificazione è questa? Tutti questi riti e salvaguardati nella legge delega in cui si prevede - altro che semplificazione! - la consacrazione della confusione che ha messo in crisi il nostro sistema processuale civile. Ecco perché il nostro voto sarà contrario, perché riteniamo che questo modo di agire non sia serio.

il gruppo della Lega Nord esprimerà un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, un disegno di legge significativamente rubricato: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile». Si tratta certamente, come da più parti è stato detto anche questa mattina pure con toni critici, di un provvedimento che contiene norme eterogenee ma aventi, tutte queste norme, una finalità univoca e comune: la modernizzazione del sistema Paese, lo sforzo di dotare il nostro Paese di strumenti più adeguati alla crescente domanda di giustizia, alla domanda di servizi per le imprese e per i cittadini, alla domanda di semplificazione della nostra pubblica amministrazione. Consentitemi una citazione, colleghi. Giuseppe Pella, economista e uomo di Governo negli anni '50 (un democristiano di altri tempi, potremmo dire), diceva: «Questo Paese non ha bisogno di aquile, ma di galline che tutti i giorni facciano l'uovo». Ritengo non sia possibile scolpire con parole più efficaci lo spirito e la *ratio* di questo provvedimento e del momento che stiamo vivendo, anche sotto il profilo della tecnica legislativa. Non possiamo, colleghi, sotto il peso incombente della crisi economica e dei gravi problemi di competitività del nostro Paese, attendere la grande riforma organica preceduta da una riflessione culturale approfondita, attendere la migliore delle riforme possibili, mentre comunque la vita scorre e pone quotidianamente problemi indifferibili. Questo provvedimento, se volete di tipo congiunturale, risponde alla necessità di dare risposte immediate; è una riforma caratterizzata da buon senso e concretezza. Questo provvedimento non promette miracoli o palingenesi, ma tenta di rabberciare qualche pezzo della sgangherata macchina giudiziaria e burocratica del nostro Paese, favorendone lo sviluppo e la competitività. Di tutte le norme che compongono questo provvedimento, per la Lega Nord significativa ed importante è senza dubbio quella contenuta nell'articolo 10 relativa ai progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale, norma che è stata migliorata grazie al nostro emendamento accolto dalle Commissioni riunite. In tale disposizione si dice che deve essere data priorità ai progetti di cooperazione allo sviluppo con i Paesi stranieri «che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime». Grazie poi al nostro emendamento a questa disposizione è stato aggiunto un ulteriore periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica». «Aiutiamoli a casa loro»: era uno slogan del nostro movimento e qualcuno ci accusa di fare politica tramite slogan. Oggi questo slogan sta diventando norma vigente. Nessuna proroga dei permessi di soggiorno degli stranieri disoccupati, ma un incentivo ai loro Paesi di provenienza per svilupparne l'economia e quindi procedere al rimpatrio degli extracomunitari disoccupati nel nostro Paese.

«Nel campo giudiziario occorrono leggine banali ma semplificatrici, una buona riorganizzazione fondata sull'informatica, giudici e personale amministrativo laboriosi, avvocati concisi». Se volete, colleghi dell'opposizione, stiamo approvando - come dice Cicala - una leggina banale, ma semplificatrice. Questa è la soluzione giusta per rendere il processo civile più efficiente e in grado di compiersi in un tempo ragionevole. Questo provvedimento contiene inoltre tre importanti deleghe: per il nuovo processo amministrativo, per la riduzione e la semplificazione dei trenta riti civili e per la mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali, favorendone la risoluzione alternativa. Conclusivamente, quindi, si tratta di un buon provvedimento, concreto e di buonsenso, che noi voteremo convintamente. Come diceva Giuseppe Pella: meglio una gallina che faccia l'uovo oggi piuttosto che un'aquila in volo nei cieli stellati delle grandi riforme.

questo provvedimento. Ma sono proprio gli interventi dei senatori Li Gotti e D'Alia che mi consentono di affrontare la questione da un altro punto di vista, più di fondo, così da illustrare argomenti generali

esso prevede poi norme sulla competitività e lo sviluppo, sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sul processo civile; questo detta il titolo del provvedimento. una violazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento: il nostro processo civile non può essere in nessun caso ridotto esclusivamente a strumento di regolamentazione Il processo civile, nel nostro Paese, ha un ampiezza molto più vasta; richiamarlo in questo modo semplificato può sviare e in qualche modo

della maggioranza e di 50 emendamenti da parte del Governo. Questo fenomeno, già gravissimo in Commissione, è proseguito e, se possibile, esaminato in scala, è anche aumentato in Aula, dove la maggioranza ha presentato 98 emendamenti

quattro deleghe al Governo; altre cinque deleghe sono contenute in emendamenti presentati ed approvati dalla maggioranza durante la discussione prima in Commissione e poi in Aula.

e dei maxiemendamenti; l'abuso dei voti di fiducia; l'abuso - ripetuto in questa legislatura in modo abnorme - dei provvedimenti cosiddetti milleproroghe; l'introduzione di questo sistema di legge "trenino" per cui al primo vagone si agganciano, man mano che proseguono i lavori parlamentari,

di esclusiva pertinenza del Parlamento e che il Governo può esercitarla soltanto in casi eccezionali, molto chiaramente sottoposti a regole precise.

alla finanziaria e lo ha fatto per introdurre un numero abnorme di modifiche ordinamentali che non riguardano solo la giustizia civile ma anche quella amministrativa (lo ricordava poco fa il senatore Li Gotti), l'ambiente, le rappresentanze consolari, la Corte dei conti (appena rimodificata in modo molto discutibile nella legge Brunetta), l'Avvocatura dello Stato, la cooperazione allo sviluppo, la tutela dell'utente, gli sprechi di carta e l'uso di Internet da parte della pubblica amministrazione, la Carta nazionale dei servizi, il risparmio energetico e persino le norme sulla bancarotta. Presidente, il Governo si è avvalso strumentalmente della rapidità dei tempi e del rigido regime di emendabilità previsto per i collegati alla legge finanziaria per realizzare a colpi di emendamenti vere e proprie riforme riforme ordinamentali alle quali il Parlamento ha sempre riservato in passato molta attenzione e che qui sono state liquidate in pochi minuti di discussione prima in Commissione sottolineo che le deleghe sono prive in gran parte dei requisiti della necessaria determinatezza, contravvenendo a quella che è una

sottolineo quello che a mio parere è il motivo più grave che ci induce a votare contro questo provvedimento: credo che nel nostro Paese sia in gioco la divisione dei poteri, in particolare il ruolo del Parlamento, in un contesto politico che ci aveva fatto sperare diversamente quando avevamo visto l'introduzione addirittura di un Ministro per la semplificazione normativa, mentre vediamo, viceversa,

Parlando dei parlamentari della maggioranza, diceva: «I parlamentari di maggioranza lamentano la loro riduzione a macchinette schiacciabottoni il cui unico contributo intellettuale consiste nel ricordarsi che il bottone verde è il secondo da sinistra e quello rosso il primo da destra». Ricordava inoltre Pera che in sostanza il presidente Berlusconi aveva detto: «ho trasformato l'Italia in una repubblica presidenziale». E spiegava

ne ha eroso la natura democratica, lo ha lasciato in sospeso ed ora lo espone persino ad avventure». Signor Presidente, prendo in prestito questa dichiarazione della perché non sto solo sollevando questioni di carattere formale e procedurale su come questa legge si è andata formando, quanto piuttosto questioni di

ci inducono a considerazioni molto gravi sulla degenerazione in atto nei rapporti tra i poteri dello Stato e nell'equilibrio tra nell'equilibrio tra i poteri stessi, fondamento della nostra democrazia parlamentare. Signor Presidente, l'Italia sta vivendo una crisi economica,finanziaria

se qualcuno pensa di risolvere la crisi aumentando i poteri del Governo,

«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile». con orgoglio e con grande senso di responsabilità l'aver compreso che vi era un nesso inscindibile tra le varie parti del provvedimento che ci accingiamo a votare Potremmo cavarcela con una battuta e limitarci a dire che le grandi pietanze sono il frutto della capacità di amalgamare tra loro ingredienti apparentemente diversi ma che, se armoniosamente fusi, rendono poi la pietanza stessa un piatto di assoluta

che esiste una connessione inscindibile tra sviluppo economico, semplificazione amministrativa e processo civile e amministrativo, nella misura in cui un Paese civile e degno di tal nome non può che avere una giustizia efficiente, anche per la necessaria tutela dei relativi diritti e della competitività complessiva del sistema Paese. Snellimento burocratico; maggiore efficienza della pubblica amministrazione; chiarezza normativa, che significa una volta per tutte comprendere ciò che una legge dice nella misura in cui abroga o sostituisce precedenti leggi, senza costringere attraverso una faticosissima sciarada a cercare affannosamente di comprendere ciò che si voleva modificare; certezza nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi, oggi sempre più strettamente interconnessi fra loro; rilancio del sistema economico. Questa è la nostra filosofia di approccio, una filosofia che - ricordo ai colleghi dell'opposizione - ha visto la maggioranza tutt'altro che prona e supina ad un testo, peraltro già largamente condivisibile, che il Governo ha portato in Aula dopo il vaglio da parte dell'altro ramo del Parlamento. lo ha letto attentamente, soppesato ed ha avanzato numerose proposte emendative che, su un impianto già sostanzialmente condivisibile, erano volte ad ottimizzarne il risultato finale, accogliendo - e non mi pare vi sia stato nessuno scadimento del dibattito parlamentare e del ruolo di questo ramo del Parlamento - numerosi e significativi emendamenti che la stessa opposizione colleghi, vi esterno una sensazione che ripetutamente ho provato e che credo abbia provato la maggior parte di noi nel corso di questo dibattito

finiscono per diventare quasi dei cavilli parlamentari. Cito un esempio che credo più di ogni altro sia illuminante al riguardo. questione sollevata in Aula ripetutamente, cioè il punto di delega per la riforma del processo amministrativo, sapendo benissimo che vi è un'interconnessione assolutamente essenziale tra la riforma del processo civile e quella del processo amministrativo se si vuole realmente che la macchina complessiva della giustizia funzioni.

per quella assoluta, inscindibile connessione che lega queste due facce di un medesimo volto; lo abbiamo fatto perché sappiamo perfettamente che, se non ci muoviamo in quella direzione, realizzeremo qualcosa che produrrà soltanto effetti parziali: e noi non vogliamo effetti parziali; con realismo e senso di responsabilità. Allora vi chiedo, colleghi dell'opposizione: non è forse indispensabile, per assicurare competitività al nostro Paese, intervenire sulle infrastrutture delle aree sottosviluppate, con adeguamenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, pubblica e privata, che oggi sono - lo dico perché un dubbio è stato sollevato - il presupposto essenziale per poter garantire competitività a quelle aree in un mondo dove l'elettronica è ormai supporto assolutamente ineliminabile? Non è forse indispensabile - ripeto - procedere alla redazione di testi normativi in modo da dare esatta e immediata contezza di ciò che si sostituisce o si abroga, rinviando in modo chiaro e integrale alle norme che si intende recepire e procedendo (perché un sistema che non ha chiarezza dal punto di vista dei riferimenti normativi è certamente di per sé stesso già farraginoso e complesso) ad una revisione ogni sette anni dei testi unici e ad una forte semplificazione legislativa? Razionalizzare e semplificare le nostre rappresentanze diplomatiche nella loro gestione non è qualcosa qualcosa che cala dall'alto del tutto improvvidamente, perché quelle rappresentanze svolgono una funzione precisa anche per ciò che riguarda l'interfaccia del sistema economico del Paese nel mondo. Dare tempi certi alla conclusione dei procedimenti amministrativi significa far sì che le nostre imprese possano lavorare con tempistiche che non siano quelle bibliche che hanno caratterizzato, troppo spesso, fasi storiche di questo Paese.

impossibilitati a svolgere le proprie attività perché, appunto, colpiti da tali patologie, con tutti i ritorni negativi che caratterizzerebbero il nostro sistema economico. Occorreva semplificare il lavoro dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti; introdurre misure di trasparenza... Grazie, Presidente. introdurre un fondo per i progetti di eccellenza in uno dei settori vitali della nostra economia, quello del turismo, rivedendo anche il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo; introdurre nuove misure di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa e del funzionamento della pubblica amministrazione; determinare tempi certi nell'erogazione dei servizi al pubblico della pubblica amministrazione; eliminare quegli sprechi cartacei, quelle montagne infinite di carte che soffocano gli uffici della nostra pubblica amministrazione; introdurre misure di risparmio energetico; e riformare, sì, significativamente il processo civile, sapendo tutti - e su questo credo che dubbio non vi sia in quest'Aula - che la riforma del processo civile non è soltanto un elemento di carattere tecnico, ma rappresenta un tassello indispensabile per ridare slancio al sistema economico del Paese. Infatti non si investe in un Paese laddove non si ha la certezza della tutela dei propri diritti. Abbiamo agito affrontando tempestivamente e convintamente quella che è ormai la parte necrotica della giustizia civile, quello che ne è il grande malato quasi terminale: il processo, la fase contenziosa, quella nella quale la tutela del diritto trova la sua più alta rappresentazione. Abbiamo operato con senso di concretezza e di responsabilità, nella consapevolezza dello stato attuale, di una montagna di cinque milioni di processi che pendono e con i quali necessariamente ci dobbiamo confrontare.

legate a una maggiore responsabilizzazione del magistrato soprattutto per quanto riguarda la durata del processo, innegabilmente oggi cozzano

questo grande malato, questa parte necrotica che in qualche modo andava sanata se non volevamo che un malato quasi terminale finisse per diventarlo Abbiamo aumentato la competenza per valore del giudice di pace; abbiamo valorizzato il principio di lealtà processuale; abbiamo semplificato la decisione della lite; i tempi per il compimento di singole attività processuali sono stati razionalizzati e accelerati; abbiamo introdotto un istituto che, sia pur contestato in quest'Aula, svolgerà una funzione acceleratrice e semplificatrice, con ritorni anche dal punto di vista economico. Infatti, così come emendato dal Gruppo di maggioranza della Commissione giustizia), l'istituto della prova testimoniale scritta significherà che decine di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori non perderanno intere giornate lavorative solo per confermare una fattura e una ricevuta fiscale. Ciò non soltanto costituisce un fatto di civiltà del diritto o di correttezza dei comportamenti processuali, ma significa far sì che questi lavoratori possano continuare a dedicarsi produttivamente alle loro attività.

ma, semplicemente, in un sistema che dà certezza delle condizioni di ammissibilità, si evita che il Supremo collegio sia soffocato da una serie infinita di questioni bagatellari, palesemente inammissibili di per sé ma che intralciano significativamente il corso e lo rivendichiamo con orgoglio - quello che è forse uno dei passaggi fondamentali della riforma del processo civile, la semplificazione dei riti, che oggi sono circa trenta e che, se il Governo opererà (e non abbiamo dubbi che lo farà) in conformità alla delega, si ridurranno a tre, a parte qualche rito speciale che comunque non faceva parte dell'impianto del processo civile strettamente inteso. Ciò significa che ne avremo eliminati ben ventitré rispetto alla dando certezza, chiarezza e tempistiche decisamente più pratiche per la tutela dei diritti. Concludendo, signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, noi voteremo con grande convinzione questo provvedimento, convinti di avere posto altre importanti tessere di quel mosaico che costituisce per noi il portato essenziale dell'essere in politica, costruire un'Italia libera, moderna, efficiente, bene amministrata, competitiva, con una giustizia degna di un Paese civile, un'Italia all'altezza delle sue tradizioni e delle grandi sfide del mondo contemporaneo.

Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per ringraziare brevemente coloro che hanno collaborato all'elaborazione, alla discussione e all'approvazione del testo: i rappresentanti del Governo, i sottosegretari Vegas e Alberti Casellati, la Presidenza del Senato, i presidenti della 1a e della 2a Commissione, senatori Vizzini

elaborato i pareri sui numerosi emendamenti, che spesso sono arrivati in tempi anche non omogenei.

il decreto‑legge in esame è volto a disciplinare i rilevanti profili in tema di quote latte, anche alla luce delle modifiche operate in sede comunitaria con particolare riferimento al nuovo livello di quota nazionale riconosciuto all'Italia, tramite un intervento di riforma su alcuni aspetti della normativa previgente, soprattutto relativamente al decreto-legge n. 49 del 2003. Si tratta, signor Presidente, di una materia che - com'è noto - ha sollevato nel corso del tempo, anche recente, profili di forte problematicità e ha suscitato tensioni e confronti in sede comunitaria e non solo, come pure atteggiamenti di aperta protesta e insoddisfazione nel contesto degli operatori del settore e degli allevatori, generando altresì contrasti ed un ampio contenzioso in sede giurisdizionale. I problemi legati alla sovrapproduzione lattiera rispetto alla quota riconosciuta all'Italia sono stati da anni una questione di difficile soluzione, che ha visto l'intervento e la mediazione di molti Governi, nel tentativo di stabilire un punto di equilibrio tra gli interessi dei produttori ed i limiti di mercato stabiliti in sede europea, con l'applicazione di sanzioni di una certa entità, che costituiscono tuttora uno dei nodi problematici di maggior rilievo. Aggiungo che il fatto di avere questo contenzioso aperto con l'Unione europea ha fortemente limitato nel tempo anche la capacità negoziale dei diversi Ministri dell'agricoltura che si sono succeduti.

che si aggiunge a quello del 2 per cento disposto dal regolamento(CE) n. 248 del 2008, che consente agli allevatori il profilarsi di una più agevole compensazione dei quantitativi in esubero produttivo.

nella prospettiva di migliorare ulteriormente la disciplina contenuta nel testo normativo in esame, proponendo altresì l'integrazione dello stesso con due articoli aggiuntivi: il primo reca un incremento della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale per la gestione dei rischi agricoli; secondo, invece, introduce una proroga delle agevolazioni previdenziali per i territori montani e le zone agricole svantaggiate. il parere della Commissione bilancio sarà determinante, per cui il relatore sin d'ora si dichiara non solo disponibile, ma interessato a valutarne le considerazioni ed eventualmente anche ad integrare o modificare le coperture previste. Passando all'illustrazione del testo, si evidenzia che l'articolo 1 detta disposizioni in materia di restituzione del prelievo e di assegnazione delle quote latte. Il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 49 del 2003 introducendo tre nuovi commi allo stesso, in base ai quali l'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota o che abbiano superato il del proprio quantitativo di riferimento individuale non si applica per il periodo 2008-2009. In un emendamento approvato dalla Commissione agricoltura, si precisa che i produttori non titolari di quote o che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale si collocano, ai fini dell'ordine di priorità per la restituzione del prelievo pagato in eccesso, dopo tutti gli altri produttori ammessi alla restituzione del predetto prelievo. ciò non è assolutamente irrilevante e voglio anche augurarmi che i manifestanti - pochi o tanti - condotti in giro per il Nord Italia

Per il periodo a decorrere dal 2009 al 2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo secondo due apposite priorità; la prima riferita alle aziende che non hanno superato il livello produttivo del periodo 2007-2008, con l'esclusione di quelle che hanno successivamente ceduto la propria quota in tutto o in parte a titolo oneroso, mentre la seconda va riferita alle aziende che realizzano un esubero contenuto entro il 6 per cento della propria quota. Le somme non restituite sono destinate ad un fondo di intervento nel settore istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 2 inserisce l'articolo 10*-bis* al citato decreto-legge n. 49 del 2003, con l'obiettivo di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dall'Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende che si trovano in una situazione strutturale di impossibilità di mantenere la produzione entro i limiti della quota e, contemporaneamente, di sopportare l'onere delle sanzioni connesse agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività - e anche per la propria sopravvivenza, vorrei aggiungere - in quanto tali aziende rappresentano quelle maggiormente produttive e vitali. La disposizione, pertanto, privilegia le aziende in maggiore difficoltà nelle assegnazioni, determinandole sulla base della situazione dell'ultima campagna lattiera conclusa e tenendo conto dei contratti di vendita di azienda e dei contratti di affitto della stessa, facendo così in modo di raggiungere l'obiettivo anche in presenza di mutamenti della conduzione. Successivamente, la stessa disposizione stabilisce i criteri di priorità delle assegnazioni verso le aziende la cui quota B è stata ridotta nel 1996, nei limiti del quantitativo effettivamente prodotto nell'ultima campagna; verso le aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al cinque per cento; infine per le aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che hanno coperto l'esubero effettivo con affitti annuali di quota. È stato approvato nel corso dell'esame in sede referente in Commissione un emendamento volto a precisare, rispetto alle aziende che hanno subito la riduzione della quota B, che l'assegnazione di quota effettuata in applicazione della disposizione in esame comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota B. Un altro emendamento assolutamente rilevante accolto dalla Commissione rimodula l'ordine di priorità previsto relativamente all'assegnazione delle quote latte, collocando in posizione equiordinata, nell'ambito del predetto ordine, le aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al cinque per cento, e le aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che nel periodo 2007-2008 abbiano coperto con affitti di quota la produzione realizzata in misura superiore al cinque per cento della quota posseduta. propone inoltre l'integrazione dell'elenco delle priorità nelle assegnazioni delle quote, di cui all'articolo 1, comma 2, con un apposito riferimento alle aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota. Questo raccogliendo le proposte di senatori, quali Santini, Zanetta, Pinzger e altri colleghi, particolarmente attenti alle problematiche dell'agricoltura e dell'allevamento in montagna. La disposizione in oggetto inoltre ricalcola il quantitativo da assegnare tenendo conto delle modifiche introdotte nell'ambito dello *Health Check* alle modalità di calcolo dell'adeguamento delle consegne in base al tenore di materia grassa, e vincola le quote assegnate a non poter essere cedute a titolo oneroso fino al 31 marzo 2015, prevedendo che in caso di cessazione dell'attività i quantitativi confluiscano nella riserva nazionale per una successiva riassegnazione. colleghi, l'articolo 2 del provvedimento dispone l'istituzione del Registro nazionale dei debiti in applicazione della normativa comunitaria in materia, nel cui contesto occorre ricordare come principi fondamentali per gli aiuti comunitari all'agricoltura sia l'obbligo da parte degli Stati membri di tutela dei fondi comunitari, almeno pari a quella dei fondi nazionali, sia l'unicità del rapporto tra produttori di attività agricola e Unione europea nell'ambito delle misure di finanziamento della politica agricola comune. L'istituzione del citato Registro è volta a garantire la massima efficienza e puntualità al recupero dei debiti maturati, sia nei confronti dell'Unione europea, sia nell'ambito della legislazione nazionale. Al Registro, istituito presso l'AGEA, sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi dovuti dai produttori agricoli, accertati dagli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, sia a titolo di prelievo supplementare sia connessi a provvidenze e aiuti agricoli erogati dalle Regioni e delle Province autonome stesse. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari e nazionali, gli organismi pagatori e le Regioni verificano presso il Registro nazionale l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero e la contabilizzazione del corrispondente importo ai fini dell'estinzione del debito, salva la possibilità riconosciuta di una soglia minima di 100 euro al netto degli interessi, al di sotto della quale è consentito agli Stati membri non procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.

dai produttori e ridurre il relativo contenzioso, evitando che il pagamento in un'unica soluzione possa determinare difficoltà economiche del debitore, tali da mettere a rischio l'effettivo recupero delle somme dovute. La finalità pertanto è quella di risolvere il problema costituito dalle ingenti somme di prelievo accumulate, in modo da contribuire alla riduzione dell'alto livello di contenzioso instaurato presso i tribunali nazionali, consentendo il versamento diluito nel tempo a quelle aziende che hanno accumulato debiti di rilevante dimensione. In questo ambito, l'articolo in questione non ammette a rateizzazione i debiti inferiori a 25.000 euro, dispone la durata massima della rateizzazione, correlata all'entità della somma dovuta, e la misura del tasso di interesse applicabile. Quindi, non stiamo parlando di nessun condono - voglio dirlo con assoluta chiarezza - ma di una rateizzazione con un tasso assolutamente di mercato. A questo proposito, si utilizza il tasso di riferimento di base previsto dalla comunicazione della Commissione dell'Unione europea sulle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Il tasso di interesse applicabile, secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del presente decreto, corrisponde mediamente al 3,6 per cento per importi tra 25.000 e 100.000 euro, con una durata della rateizzazione non superiore a dieci anni; al 4,6 per cento per importi maggiori di 100.000 euro e non superiori ai 300.000, con una durata non superiore a venti il 5,6 per cento per importi maggiori di 300.000 euro, con durata non superiore a trenta anni. La materia della rateizzazione dei debiti è oggetto altresì dell'articolo 4, il quale detta disposizioni integrative a quelle dell'articolo precedente definendo i passaggi procedurali finalizzati alla rateizzazione. La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha approvato un emendamento in cui si precisa, in riferimento alla disposizione prevista al comma 1 - relativa all'obbligo per l'AGEA di inoltrare, entro 45 giorni, un'intimazione a ciascun debitore per le somme esigibili che sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. Un altro elemento accolto dalla Commissione dispone che tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento inoltrate, al fine di evitare che l'inoppugnabilità degli atti precedentemente notificati possa venir meno a seguito dell'invio di una nuova intimazione, suscettibile di riaprire i termini per l'impugnativa in sede giurisdizionale. Faccio notare, cari colleghi, che questi due emendamenti potrebbero essere definiti, molto sbrigativamente ma anche esattamente, emendamenti anti-furbetti. Qualcuno nei giorni scorsi ha parlato di intento del Governo di proteggere i furbetti: ebbene, non è così e i due emendamenti appena citati sono proprio volti ad evitare che a qualcuno possa venire in mente di fare ancora il furbetto. La Commissione ha poi proposto un'integrazione del testo, con la quale si dispone, in riferimento alla norma contenuta al comma 4, che i debiti di prelievo supplementare che si rendono successivamente esigibili devono essere riferiti necessariamente ai periodi precedenti al 2008-2009. In particolare, l'articolo in questione prevede che l'istruttoria individuale delle richieste presentate sia affidata ad un apposito commissario straordinario, nominato fino al 31 dicembre 2010, che avvalendosi del supporto dei competenti uffici dell'AGEA assegna le quote aggiuntive concesse all'Italia, determina l'accoglimento o meno della richiesta presentata e, in caso di accoglimento, le modalità di rateizzazione. Tali competenze passano all'AGEA dal 1° gennaio 2011. Relativamente all'istituzione di un commissario straordinario, prevista al comma 5 dell'articolo 4, si è ritenuto necessario introdurre, con apposito emendamento approvato dalla Commissione, una nuova prescrizione in base alla quale si dispone che tale incarico venga attribuito a un soggetto scelto tra i dirigenti del Ministero e delle società controllate, in modo tale da evitare che tale organo si collochi al di fuori del contesto organizzativo del Dipartimento. Anche questo, voglio ricordarlo, è un emendamento di garanzia, per evitare che magari vengano effettuate nomine di commissari strane o stravaganti, che non fanno riferimento all'amministrazione delle politiche agricole. La Commissione che ho l'onore di presiedere Presidente, una modifica con la quale si stabilisce che per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. Ed anche questo non è poco. Un altro emendamento accolto dalla Commissione, che prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione per il mancato pagamento anche di una sola rata, elimina qualsivoglia eccezione rispetto a tale decadenza, in modo tale da evitare che l'efficacia deterrente della disposizione in questione venga vanificata attraverso una serie di deroghe introdotte in via regolamentare. Viene poi previsto, attraverso un apposito emendamento accolto dalla Commissione, al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti connessi al regime delle quote latte, che gli incarichi dirigenziali dell'AGEA conferiti con contratti a tempo determinato siano rinnovabili due volte anziché una sola volta, come previsto dalla normativa vigente. La disposizione prevede altresì la revoca delle quote assegnate per le ipotesi di mancato pagamento del prelievo latte, di omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine, rigetto della richiesta di rateizzazione, di rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente della proposta di rateizzazione formulata dal commissario straordinario. inoltre che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione ed in quelle di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata. L'articolo 5 stabilisce che le disposizioni degli articoli 3 e 4 in materia di rateizzazione dei debiti siano applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009. L'articolo 6, infine, prevede che le somme versate dai produttori di latte affluiscano ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario: alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 ed a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. che alle misure di accesso al credito, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è assegnata la somma di 25 milioni di euro, da destinare prioritariamente ai produttori che abbiano acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003, convertito dalla legge n. 119 del 30 maggio 2003. maggio 2003. È previsto tra l'altro un subemendamento del relatore, già presentato, che porterebbe tale somma da 25 a 35 milioni. È chiaro che se applichiamo un coefficiente di moltiplicazione

tra l'altro da aggiungere al cofinanziamento di privati; quindi si andrebbe ad attivare un fondo di 700 milioni di euro. Qualche giorno fa il Ministro e tutti quanti noi abbiamo ascoltato la richiesta reiterata di 700, 500, 300 milioni, tra l'altro vi sono anche numerosi emendamenti al riguardo; ebbene proprio questo viene garantito. Faccio anche presente che se il decreto-legge avesse previsto effettivamente 500 milioni, moltiplicati per dieci avrebbero dato vita a cinque miliardi, che poi moltiplicati per due per il cofinanziamento sarebbero stati dieci miliardi di euro per quanti hanno acquistato le quote latte, cosa che francamente mi sembrerebbe un po' eccessiva rispetto alle esigenze generali del comparto dell'agricoltura in questo momento. La Commissione propone inoltre l'introduzione di un articolo aggiuntivo al decreto in esame, ossia l'articolo 6-*bis*, relativo alla gestione dei rischi agricoli (come dicevo in precedenza), finalizzato ad incrementare di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 il Fondo di solidarietà nazionale. Infine, con apposito emendamento accolto dalla Commissione, si propone la proroga al 31 dicembre (o eventualmente al 30 giugno, seguendo l'impostazione del Presidente della

sono assolutamente convinto che il Ministro abbia fatto un eccellente lavoro di forte rivendicazione a Bruxelles. Con assoluta determinazione e con consapevolezza dei gravi problemi di tutta l'agricoltura italiana, non solo del comparto lattiero, ha portato a casa un risultato estremamente importante. Il presidente Berlusconi in prima persona ha garantito al Ministro dell'agricoltura un appoggio, una copertura, la più autorevole possibile, presso il Presidente della Commissione europea e penso che il Ministro ne sia assolutamente consapevole. Quindi è stato raggiunto un risultato estremamente rilevante. È evidente che a questo punto occorre distribuire equamente le nuove quote ottenute e che è opportuno procedere ad una rateizzazione equa; è evidente, insomma, che occorre cercare di garantire un po' di serenità a questo comparto, superare le difficoltà, superare i contenziosi e le proteste che si sono avute negli anni che hanno dato luogo anche ad episodi estremamente spiacevoli, e guardare con maggiore decisione e maggiore serenità alle nuove partite, alle nuove battaglie che si dovranno combattere a livello comunitario e soprattutto internazionale per difendere l'agricoltura italiana.

Signor Presidente, com'è noto il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, reca una serie di misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. In altri termini, le due questioni che il provvedimento in esame contiene riguardano, da un lato la necessità di assicurare l'assegnazione del quantitativo nazionale di latte ai produttori e, dall'altro, di assicurare la rateizzazione dei debiti contratti dagli allevatori relativamente alle cosiddette quote latte. Dal nostro punto di vista, questa proposta presenta alcuni evidenti profili di incostituzionalità. Il primo è noto, ovviamente, e riguarda la violazione dell'articolo 77 della Costituzione sotto il profilo della

non emerge alcuna circostanza oggettiva a supporto dei motivi di necessità ed urgenza, ma - com'è noto - il presupposto dell'urgenza, che è autonomamente giustiziabile, è facile da verificare in quanto consiste nella inevitabilità ed improrogabilità della norma da adottare per risolvere una situazione di carattere straordinario. Nel caso di specie tale presupposto manca del tutto, posto che si tratta di un intervento non giustificato da alcuna urgenza, anche in considerazione del fatto che in Italia vi è un problema strutturale di carenza delle quote latte, confermato dall'elevato contenzioso instaurato negli ultimi anni innanzi ai tribunali nazionali avverso le sanzioni che sono state via via comminate per gli eccessi di produzione non autorizzati. Manca pertanto tale presupposto ed al riguardo, come è noto, la stessa Corte costituzionale anche di recente con la sentenza n. 171 del 2007

viene viziato il decreto-legge e che il vizio si estende al procedimento e, quindi, alla relativa legge di conversione. Per quanto riguarda il provvedimento che siamo chiamati oggi ad esaminare, più nello specifico - dal nostro punto di vista - la violazione e la dedotta carenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione va riferita agli articoli 3 e 4 del decreto, che perseguono l'obiettivo di garantire il recupero degli importi dovuti dai produttori con modalità sostenibili. Si tratta di un intervento ordinario, strutturale, connesso peraltro alla esigenza di recuperare gli importi già versati dall'Italia all'Unione europea.

(che, come è noto, sancisce i princìpi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) e 41 della Costituzione, che contiene l'enunciazione del principio della libertà di iniziativa economica e privata. parola, infatti, in maniera del tutto irrazionale introducendo disposizioni di favore per coloro i quali hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, accumulando debiti di dimensioni rilevanti ed alterando quindi il sistema della libera concorrenza fra i produttori, agevola non coloro che non coloro che hanno rispettato la legge e che si sono messi in regola ma coloro i quali la legge non l'hanno rispettata e attribuisce all'amministrazione una funzione pubblica discriminatoria nel rapporto fra diversi soggetti che operano nello stesso mercato. Più precisamente, l'articolo 3 del una sanatoria a favore dei produttori che nel corso degli ultimi anni hanno sforato le quote di produzione loro assegnate consentendo di rateizzare i debiti iscritti nel Registro nazionale dei debiti Tale norma risulta del tutto irrazionale anche in considerazione del fatto che introduce una evidente disparità di trattamento rispetto ai produttori che, viceversa, in maniera assolutamente diligente e rispettosa della norma seppure in una congiuntura di mercato non favorevole, hanno provveduto al versamento delle somme dovute. il decreto in parola presenta un complesso di interventi in favore di tutti coloro che fino ad oggi hanno operato al di fuori della legge, prevedendo addirittura discriminazioni nei confronti della grande maggioranza degli allevatori che, con enormi sacrifici, in questi anni hanno rispettato le regole. evidente la ingiustificata differenziazione tra la disciplina introdotta in favore di questi produttori ed una disciplina che invece penalizza quei produttori che hanno scelto di operare legittimamente e regolarmente. Da ultimo, signor Presidente, appare del tutto irrazionale anche la scelta di favorire, nell'assegnazione delle nuove quote disponibili, i cosiddetti grandi splafonatori, splafonatori, soggetti privilegiati nell'assegnazione delle quote aggiuntive, che non sono tenuti neppure a rinunciare al contenzioso aperto contro lo Stato per temporeggiare sul pagamento delle multe, mettendo sostanzialmente in coda coloro che hanno rispettato i dettami della legge 30 maggio 2003, n. 119.

alla tutela di altri furbetti: dalla tutela dei furbetti del quartierino, alla tutela dei furbetti del latticino. Io credo che questo non sia consentito, perché alla fine ciò che si determina è la penalizzazione di un comparto importante, che gran parte del prodotto interno lordo del nostro Paese e che ha bisogno, secondo me, di regole che siano sottratte al voto di scambio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente voteremo negativamente rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dal collega D'Alia,

ogni volta nell'ambito delle questioni pregiudiziali viene sollevata la mancanza dei presupposti richiesti per la decretazione d'urgenza. L'interpretazione corretta che ne ha dato la Corte valorizza invece anche la discrezionalità politica del Governo in merito e, quindi, valorizza l'oggettiva urgenza di provvedere. Correttamente, nel preambolo del decreto-legge, si dice testualmente: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile».

la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, basata sull'assunto di una discriminazione rispetto a coloro che in passato hanno sostenuto sforzi per rispettare il regime delle quote latte, anche in questo caso la questione pregiudiziale omette alcuni passaggi. L'accesso ai benefici, alle nuove assegnazioni e alla rateizzazione recata dal presente decreto‑legge è sempre e comunque onerosa,

Quindi, il provvedimento in esame non è assolutamente da considerare un provvedimento discriminatorio nei confronti di chi in passato ha rispettato il regime delle quote latte e non è assolutamente da considerare una sanatoria,

una concreta possibilità di regolarizzazione a titolo oneroso; vogliamo ribadire questo aspetto: a titolo oneroso. Si tratta di un provvedimento

Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della questione pregiudiziale proposta dal senatore D'Alia. Tale questione opportunamente evidenzia l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, per le ragioni che abbiamo ascoltato, e sottolinea i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento dell'enorme rateizzazione concessa ad alcuni produttori con gli articoli 3 e 6

che hanno rispettato le regole e coloro che non hanno rispettato le regole, e che determina anche una distorsione delle regole della concorrenza tra chi ha pagato, pur in presenza di difficoltà

non abbiamo voluto presentare una questione sospensiva perché conosciamo la prassi sin qui seguita. Si tratta di questo.

perché, in modo del tutto fantasioso e innovativo, la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto che allungare i pagamenti fino a trenta anni allungare i pagamenti fino a trenta anni di somme peraltro già sborsate dallo Stato per mezzo dell'AGEA all'Unione europea

in attesa di verificare cosa il Governo risponderà sulla questione, vorrei sollevare il problema, che in altra circostanza abbiamo seppur incidentalmente fatto

copertura finanziaria investono l'aspetto centrale del provvedimento stesso, quindi anche questioni di merito e di sostenibilità della disposizione normativa oggetto del disegno di legge. che conosco bene la prassi in base alla quale la mancanza del parere della 5a Commissione non preclude lo svolgimento della discussione generale, ma soltanto l'inizio delle votazioni sugli emendamenti

rivisitata e riesaminata la prassi applicativa delle norme regolamentari, per esempio, sul regime dell'ammissibilità degli emendamenti, dei decreti-legge e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, come è accaduto nei nei giorni scorsi. Ritengo - e in questo senso la sollecito - che sarebbe opportuno stabilire che, allorquando la 5a Commissione non ha completato l'esame dei provvedimenti sotto il profilo della copertura, che però investe la sostenibilità della norma di cui si discute, bisognerebbe far seguire la discussione generale all'espressione del parere

Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, con il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, il Governo introduce un insieme di norme in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. un decreto-legge che, lo voglio ricordare, ha origine dal negoziato sulla verifica dello stato di salute

con il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, il Governo introduce un insieme di norme in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. un decreto-legge che, lo voglio ricordare, ha origine dal negoziato sulla verifica dello stato di salute della politica agricola comunitaria conclusosi a Bruxelles lo scorso 20 novembre, un negoziato che, per lo specifico tema delle quote latte, ha assegnato all'Italia un ampliamento delle quote del 5 per cento, come per tutti gli altri partner europei, con l'unica differenza che al nostro Paese è stato concesso di farlo in maniera anticipata e con il preciso obiettivo di stabilizzare il mercato sanando le irregolarità di cui sono stati protagonisti alcuni produttori italiani. Il Governo ha parlato di un risultato storico, ma non si capisce per chi e perché. Se questo è un risultato storico, cosa è stato allora quello del 1999, quando soltanto l'Italia riuscì a portare a casa un aumento di circa 600.000 tonnellate di quote latte all'interno di Agenda 2000? Al di la dei paragoni, è importante evidenziare che la politica degli annunci non giova al Paese. L'agricoltura italiana, e nello specifico il settore lattiero-caseario, affronta oggi uno scenario fatto di mille difficoltà, amplificate dalle sue deficienze strutturali e organizzative e dalla crisi internazionale su cui occorre riflettere. Alla luce dei contenuti del decreto-legge varato dal Governo sembrerebbe piuttosto che il risultato sia stato storico non tanto per il comparto, quanto per quei produttori che fino ad oggi hanno trasgredito le regole, a beffa di quelli che invece le hanno sempre rispettate.

Inizialmente, dopo i cicli di audizione che si sono svolti sia al Senato che alla Camera, avevamo anche apprezzato la disponibilità del Governo a modificare i contenuti del provvedimento. Purtroppo però, come è accaduto sin dall'inizio di questa legislatura, ancora una volta non sono state mantenute Le principali proposte di modifica presentate in Commissione agricoltura dai senatori del Gruppo PD - un pacchetto di emendamenti particolarmente orientato a favore di coloro i quali nel corso degli anni hanno rispettato le regole ed agito nella legalità, condiviso dal mondo produttivo e da tutte le Regioni - sono state fino ad oggi respinte dal Governo. Ed ora, brevemente, vorrei chiarire in maniera dettagliata, seppur sintetica, la nostra posizione, perché noi non facciamo disinformazione e non diciamo bugie. All'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in discussione, abbiamo chiesto di invertire l'ordine di priorità di assegnazione delle quote, portando gli affittuari al secondo posto e gli splafonatori al terzo. Il Governo ha ritenuto opportuno accorpare in unica categoria gli affittuari e gli splafonatori. Un aggiustamento che non accontenta nessuno ed è, al tempo stesso, iniquo. Infatti, dai risultati dei la quota di tutti gli splafonatori e degli affittuari risulterebbe coperta al 60 per cento rispetto al fabbisogno reale. Ricordo, onorevoli colleghi, che se le produzioni non fossero state coperte da affitti, sarebbero rientrate fra gli esuberi. L'affitto è una manifestazione della volontà del rispetto delle regole e deve essere prioritario nell'assegnazione delle quote rispetto a chi le regole, invece, le ha infrante. Sempre all'articolo 1 abbiamo proposto, ancora una volta senza ottenere riscontri positivi, la soppressione del comma 1 sia perché inserisce regole con effetto retroattivo (campagna 2008-2009) sia per evitare che chi ha splafonato oltre il 6 per cento della propria quota produttiva, pur essendo in regola con i versamenti delle multe, si veda escluso dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso.

e, al tempo stesso, non ostacolare la partenza del processo di assegnazione delle nuove quote prevista per il 1° aprile, abbiamo presentato un emendamento per far confluire in riserva nazionale le assegnazioni previste per i produttori con prelievo supplementare non versato fino alla definizione del procedimento di rateizzazione. Signora Presidente, le quote da assegnare in riserva nazionale (prima, non dopo le adesioni alla rateizzazione) devono riguardare tutti i produttori con prelievo non versato e non solo quelli con debiti esigibili, come indicato in un emendamento del Governo presentato all'ultimo momento nella giornata di ieri nel tentativo, non riuscito per altro, di confondere le idee. All'articolo 3, comma 2, abbiamo presentato un emendamento che contenesse la rateizzazione in un massimo di 20 anni.

un comma aggiuntivo affinché i soggetti che aderiscono alla rateizzazione delle multe pregresse, così come previsto dalla citata legge n. 119, debbano rinunciare espressamente ad ogni azione giudiziaria intrapresa. Il Governo ha ritenuto che non fosse un aggiustamento necessario decidendo, al contrario, di schierarsi a favore degli splafonatori che non hanno versato le multe. Sempre all'articolo 4 del disegno di legge in esame

pagamento di almeno una rata di multe pregresse e, al tempo stesso, l'AGEA possa trattenere in via preventiva i premi PAC di spettanza del debitore versamento delle singole rate. Ebbene, anche qui il Governo ci ha dato un "contentino" accogliendo esclusivamente la proposta che prevede di trattenere gli aiuti PAC, ma solo sul pagamento della prima rata della multa, che tra l'altro non dovrà essere versata in anticipo. che il fondo dedicato ai produttori di latte che hanno rispettato le regole deve essere assolutamente dedicato a coloro i quali le regole le hanno rispettate e che hanno pagato, salate, le quote degli anni precedenti.

ma certamente non è sufficiente, così come non sono sufficienti gli emendamenti presentati ieri sera. Stiamo lavorando per dare una risposta agli allevatori onesti che hanno rispettato le regole.

sostenendo)? Abbiamo davvero toccato un punto delicato, perché le Regioni sono state totalmente escluse e, non a caso, all'unanimità esse hanno espresso un parere contrario alla proposta del Governo. Al contrario il Partito Democratico, a nome del quale ho preso la parola, ritiene indispensabile che coloro i quali hanno continuato a produrre latte ignorando la legge paghino prima gli arretrati e poi ricevano le nuove una proposta trasparente e all'insegna dell'onestà, contenuta negli emendamenti presentati dai colleghi senatori del PD della Commissione agricoltura e che si spera possa essere accolta in quest'Aula.

si consumavano le proteste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria. Ciò non ha prodotto significativi miglioramenti del testo al nostro esame, nonostante il ministro Zaia abbia più volte dichiarato di essere ad accogliere alcune correzioni al decreto sulla base delle richieste avanzate in Parlamento. In realtà, tutte le principali richieste avanzate in Commissione agricoltura dall'opposizione, condivise dal mondo produttivo, dalle associazioni di categoria e dalle Regioni sono state respinte dal Governo. Le uniche parziali modifiche accolte dal ministro Zaia non risolvono le problematiche sollevate a gran voce in questi giorni dagli operatori del settore, lasciando al contrario invariate le norme più critiche di questo decreto-legge, come ad esempio il famoso comma 1 dell'articolo 1 relativo ai nuovi criteri di compensazione nazionale o di restituzione del prelievo versato in eccesso, che penalizzano tutti coloro che fino ad oggi hanno sempre operato nel rispetto della legislazione vigente.

questo settore e lo facciamo con molta attenzione, perché riteniamo - l'ho sempre detto - che questo è l'unico comparto che ci dà la possibilità di riportare lo sviluppo economico e occupazionale nel Paese. Dobbiamo essere grati a questa

Il decreto-legge al nostro esame, in sostanza, sancisce la rateizzazione delle multe pregresse e la ripartizione delle nuove quote assegnate all'Italia. Siamo costretti a pronunciare un giudizio molto critico, come dicevo prima, sul decreto-legge, in particolare perché il ministro Zaia, con questo provvedimento, ha deciso di tenersi in portafoglio le nuove quote, che quindi non verranno ripartite tra le Regioni (alla faccia del federalismo!), come prevedeva la legge n. 119 del 2003. Sarà quindi lo Stato a decidere in merito alla distribuzione delle quote. Le nuove quote saranno assegnate in parte ai produttori responsabili delle eccedenze ed in parte agli altri produttori. Nel decreto, inoltre, si prevede l'inserimento delle zone svantaggiate, accanto a quelle di pianura, quali destinatarie prioritarie delle ulteriori quote latte assegnate all'Italia dall'Unione europea. Se sulla distribuzione delle quote sarà lo Stato a decidere, a proposito di dilazione e pagamento delle multe la situazione che emerge appare più chiara. La questione interessa 8.404 aziende, di cui 4.264 ancora in attività, mentre 1.500 sono quelle che devono ancora pagare le multe accumulate nell'ultima campagna lattiera. Il totale di questo contenzioso raggiunge 1.671 miliardi di euro, il totale delle multe in 24 anni ammonta a 3 miliardi, mentre complessivamente tutta la partita delle quote latte è costata al Paese 9 miliardi di euro. Il decreto-legge chiarisce che l'esigibilità delle multe avverrà a mano a mano che arriveranno le sentenze relative ai vari contenziosi e i pagamenti andranno automaticamente in rateizzazione. Le multe comunque, secondo quanto prevede il decreto-legge, verranno rateizzate a titolo oneroso, con un interesse importante, anche eccessivo per i produttori, che può arrivare fino al 7 per cento, nonché con limiti temporali già stabiliti a livello europeo per il pagamento della multa. Ho visto però qualche nuovo emendamento

degli allevatori. Secondo il Gruppo dell'Italia dei Valori, fra i punti più controversi del decreto-legge al nostro esame figura proprio l'articolo 1, comma 1, che prevede la riammissione alla compensazione nazionale della campagna lattiera in corso, che nulla ha a che fare con la distribuzione delle quote aggiuntive autorizzata da Bruxelles degli allevatori privi di quota e di quelli che hanno prodotto più del doppio della quota assegnata. Questo significa ridurre drasticamente le possibilità di compensazione per coloro che rispettano le normative. Degli articoli successivi si conferma che le quote aggiuntive vengono assegnate soprattutto ai grandi splafonatori, mettendo in coda coloro che hanno pagato per avere le quote necessarie in affitto, limitando la restituzione della quota "B" tagliata al solo quantitativo prodotto in esubero, mentre i piccoli splafonatori vengono addirittura esclusi dall'assegnazione. Circa poi il famoso fondo finanziato con i versamenti di coloro che si metteranno in regola, si tratta in realtà di pochissime briciole, poiché i fondi

Come preannunciato, inoltre, non si chiede la rinuncia al contenzioso, ma al contrario si introducono ulteriori elementi controversi, che potranno incrementare il ricorso ai tribunali. come già accennavo, viene disconosciuto l'operato delle Regioni, alle quali si riserva il ruolo di postini, nel senso che devono limitarsi a comunicare le assegnazioni alle aziende. In conclusione, signor Ministro, al di là dei criticabili contenuti del decreto-legge che questo ramo del Parlamento sta per approvare, francamente in questo momento la mia preoccupazione è rivolta maggiormente verso il prezzo del latte che sta precipitando e verso gli industriali,

Questi sono i veri problemi: si utilizza latte estero, che non viene immesso nel mercato di quel Paese, per non abbassarne i prezzi interni, e viene portato sul nostro Paese a prezzi ridicoli. Questo non è un mercato equilibrato e normale:

Lo sa che alcune industrie comprano il latte magro, lo ricostituiscono e poi lo fanno entrare nella filiera del latte? L'aumento di quota in questo periodo causerà un eccesso di offerta ed un conseguente crollo del prezzo del latte alla stalla, che si allineerà ai valori di Germania (30 centesimi al litro) e Francia (29). Il Ministro con questo aumento riuscirà a non far chiudere 1.500 stalle di allevatori irregolari. Il crollo del valore delle quote latte, che andranno quasi a zero, e la riduzione del prezzo del latte, in compenso, causeranno un crollo dei redditi di tutti gli agricoltori: credo che per molti di loro sarà molto duro continuare ad operare se il prezzo scenderà a tali livelli. livelli. Gli operatori del settore avrebbero desiderato altri interventi, basati soprattutto sul rispetto della legge esistente, la famosa n. 119 del 2003, proposta dall'allora ministro Alemanno e approvata in modo *bipartisan* in Parlamento. Questo vuole dimostrare che l'opposizione non dice solo no, ma a volte riesce in modo costruttivo a produrre buone leggi. Quando parlo di rispetto della legge n. 119 intendo dire di assegnare in tempi rapidi l'aumento di quota agli aventi diritto. Ovviamente le stalle irregolari dovranno saldare la situazione pregressa anche con rateizzazioni e poi ottenere la loro parte di aumento, ma nessuno dei produttori regolari vuole concedere regali a chi fino a ieri gli ha fatto una concorrenza sleale.

attraverso la propria rappresentanza parlamentare in Commissione agricoltura del Senato e della Camera ha partecipato, su invito del ministro Luca Zaia, a più di un confronto sui contenuti del decreto sulle quote rassegnando poi per iscritto una posizione ben precisa, articolata in sei punti, così intendendo conferire un apporto estremamente costruttivo e interpretando correttamente e serenamente le ragionevoli aspettative del settore interessato.

è stato appena detto, fu votata da larga parte del Parlamento. Auspicammo particolarmente che di quella legge si cogliesse almeno l'importanza del ruolo che essa affida alle Regioni, quali organi deputati all'amministrazione delle È invero abbastanza strano che un Governo tanto orientato sul federalismo non valorizzi tale aspetto, e in ogni caso abbia escluso le Regioni da un preventivo confronto su un tema così avvertito. È rimasta invece forte nell'Esecutivo la tentazione di accentrare nelle proprie mani incombenze squisitamente gestionali che già oggi, a legislazione vigente, non dovrebbe assumere. Più strano ancora appare tutto ciò in relazione all'appartenenza politica dell'attuale titolare del Ministero delle politiche agricole. Tuttavia, le premesse lasciavano intendere che vi fosse una reale volontà

non si tratta soltanto di una chiusura politica al maggior partito di opposizione, che - è bene saperlo - proseguirà nel suo impegno senza sosta e senza indietreggiamenti, di un sonoro schiaffo alla stragrande maggioranza dei produttori, rispettosa delle regole, che ha operato nella legalità ed in cambio riceve una forte penalizzazione dal Governo.

che non ha trovato ascolto. Non solo, ma in questi giorni si è maldestramente tentato di svilire le manifestazioni di civile protesta e le vibrate reazioni delle categorie interessate, al livello di una volgare strumentalizzazione. Non è così! Il mondo agricolo non si sarebbe prestato, se mai qualcuno avesse tentato di utilizzarne la buona fede ed il sacrificio che quotidianamente affronta. Ho girato molto in questo periodo ed ho potuto percepire con nettezza la distanza vera e profonda che, anche nel settore primario, separa il Paese reale dal Paese legale. La mobilitazione nella pianura padana, così come in vaste zone dell'Italia settentrionale, è vera ed avvertita. I presìdi lungo i principali assi viari sono lì da settimane: spesso sono frequentati ed animati da donne ed uomini che magari hanno votato alle scorse elezioni politiche per i partiti della maggioranza, e che oggi sentono tradita la fiducia che in essi avevano riposto. Come pure devo dire di avere registrato - rispetto alle posizioni permissive, addirittura elogiative, che la più grande organizzazione professionale del mondo agricolo ha assunto in sede nazionale - una evidente divaricazione di significative espressioni dei suoi quadri periferici nel giudizio sul decreto quote latte.

trovino oggi ospitalità all'interno di un contenitore improprio quale quello del decreto sulle quote latte. Va detto però - e me lo si deve consentire che lo strumento dentro il quale sono collocati tali provvedimenti non è adeguato: abbiamo avuto occasioni diverse per poter dare risposte. Mi sembra che ci sia invece un tentativo di azzardare una sorta di compensazione sul piano del consenso del mondo agricolo. Non intervengo, e concludo, nel merito delle questioni relative al decreto perché già trattate in modo esauriente da par suo

che, al contrario, prevede la rinuncia al contenzioso prima di accedere al beneficio e sarebbe perciò quanto mai utile un adeguato approfondimento al riguardo. Mi limito in conclusione a dire che le risorse assegnate a sostegno del settore lattiero-caseario sono insufficienti rispetto alle quote acquistate e, soprattutto, penalizzano chi ha sempre operato nella legalità. II PD è vicino ai tantissimi allevatori che stanno legittimamente manifestando

di capire che questo decreto sulle quote latte è un ingiusto regalo a quei pochi che hanno guadagnato sulle spalle degli onesti, una sorta di condono mascherato a favore di chi ha agito nell'illegalità.

siamo consapevoli di quanto sia indispensabile chiudere questo doloroso capitolo della storia dell'agricoltura italiana, che è costata in termini economici, di immagine e di credibilità del Paese, per concentrarsi finalmente sulla soluzione dei problemi vari, problemi vari, ma anche veri del settore lattiero-caseario, attanagliato dall'azzeramento della redditività e sempre più stretto dai vincoli ambientali, sanitari ed urbanistici. La conclusione cui ci porta il decreto-legge e le proposte emendative presentate in Commissione agricoltura nonché quelle presentate *in extremis* dal Governo non rispondono appieno alle aspettative del comparto interessato. Aspettative di una piena tutela della legalità, della giustizia e dell'equità avanzate dai tanti allevatori onesti che hanno investito ingenti somme per acquisire le quote produttive, gravando così le proprie imprese di oneri finanziari, oggi bisognosi di sollievo. In tal senso sosteniamo ed appoggiamo le misure volte a dotare il Fondo di risorse finanziarie adeguate, a ridurre il peso delle garanzie delle aziende che hanno agito nel rispetto delle regole e nella correttezza. La sola prospettiva di premiare chi ha perseguito comportamenti illegali per 25 anni nella irrisione della stragrande maggioranza degli allevatori onesti sarebbe una beffa, la risposta più sbagliata che il Governo possa dare al Paese, dal quale si eleva una diffusa domanda di legalità. Dare una risposta sbagliata oggi non solo nuoce alla credibilità del Governo, ma investe anche quella del Parlamento e delle istituzioni tutte. Il Governo ed il ministro Zaia dimostrino con i fatti che le cose non stanno così, che non ci sono elementi di iniquità nell'assegnazione delle quote aggiuntive, che la rinuncia ai contenziosi è specchio di una legalità recuperata da quanti per troppi anni l'hanno aggirata. Abbiamo raccolto la preoccupazione, ancora diffusa tra gli operatori e i conoscitori del settore, che ad antiche furbizie se ne aggiungano delle nuove e che i vincoli inseriti nelle procedure di regolarizzazione delle multe pregresse non siano tali da evitare reiterati tentativi di elusione. Proprio per questo, nel momento in cui si chiedono sacrifici e rigore al Paese bisogna dare messaggi e regole in coerenza. Questo provvedimento ne può essere un utile esempio ed il pronunciamento del Senato ne porterà tutta la responsabilità. Il percorso di condivisione che c'era stato chiesto aveva trovato nei componenti della Commissione agricoltura del Partito Democratico un appoggio convinto e leale che purtroppo è stato via via disatteso da una chiusura sui punti fondanti del Partito Democratico, richiamati poc'anzi dal collega Andria. Noi di questo decreto-legge cogliamo anche gli aspetti positivi,

Signora Presidente, il poco tempo concessomi mi induce ad entrare rapidamente nel tema che intendo trattare, quello dell'agricoltura di montagna e dei riflessi che questa grande riforma può avere anche su di essa. Del resto, i temi generali, gli aspetti importantissimi e storici di tale riforma, sono stati già tracciati, con la nota perizia, dal nostro relatore ed altri saranno evidenziati in fase di dichiarazione di voto dal senatore Sanciu, nostro Capogruppo

di un dibattito e di un confronto molto difficile e delicato, di concedere un piccolo spazio di attenzione e considerazione anche alla specificità della montagna. Questo è avvenuto non soltanto con pacche sulle spalle o espressioni demagogiche, ma con l'accettazione di un paio di emendamenti che hanno consentito di inserire - lo ha ricordato il relatore poco fa - nell'importante articolo 10-*bis*, dove si parla di assegnazione di quote, al comma 4, lettere *b)*

l'Europa avrebbe finito per mettere un palo fra le ruote anche a tutto il resto. Quindi, abbiamo rinunciato a questa idea che tuttavia, magari in sede di discussione di emendamenti, ricorderò per rendere onore e omaggio ai protagonisti di tale emendamento, che sono i giovani

di continuità, di presenza, di speranza che qualcuno possa rimanere in quelle zone. Signor Ministro, le dico queste parole, che potrebbero apparire anche ispirate a piaggeria,

la soma è stata un po' raddrizzata; ora il testo incontra il favore anche di questa piccola categoria di allevatori. Gli allevatori di montagna e i giovani, in modo particolare,

è garanzia assoluta per poter riequilibrare quegli scossoni, quelle difficoltà che per questo tipo di allevatori sono pane quotidiano. Quando si registrano produzioni minori o inferiori in montagna non dipende dal capriccio di chi è coltivatore o allevatore in ma da eventi esterni che nessuno può controllare. Quindi non si sta parlando di nessun furbetto, ma di gente seria, che ha deciso con una scelta precisa di rimanere a lavorare, a vivere e a cercare un reddito adeguato laddove è più difficile ottenerlo. queste piccole attenzioni, queste misure che riguardano una minoranza dei nostri agricoltori contribuiscono a dare speranza e a lottare contro il pericolo maggiore che esiste in montagna, ossia l'esodo. Rimanere lassù, spesso con un'attività agricola prevalente, è il punto di partenza per garantire quella multifunzionalità che spesso significa, per le zone di montagna, salvezza generale dell'ambiente, delle condizioni di vita e di lavoro e di molte altre attività parallele. Quindi rinnovo il compiacimento e chiaramente chiederò al mio coordinatore di esprimere un voto favorevole anche per questi dettagli, accanto ai molti altri motivi positivi che egli ricorderà. link apre una nuova finestra") *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, siamo chiamati in queste ore a pronunciarci sul decreto in materia di produzione lattiera e di rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, proprio nel momento in cui varie manifestazioni di protesta e di insoddisfazione sono cresciute e si stanno diffondendo in diverse zone del Paese. Per riportare la discussione nei binari della verità e del merito, rispetto alle reazioni scomposte cui invece abbiamo assistito negli ultimi giorni (mi riferisco, ad esempio, al volgare e personale attacco al presidente lombardo di Confagricoltura, così come agli agricoltori riuniti in presidio a Parma), credo sia corretto e doveroso ripercorrere le settimane trascorse dall'emanazione del decreto ad oggi. Il provvedimento è nato con l'obiettivo di chiudere un contenzioso che si sta trascinando da circa 25 anni, un contenzioso costato agli italiani circa 2,5 miliardi di euro versati all'Unione europea. Su questo obiettivo, lei potrà dare atto, signor Ministro, che come Partito Democratico abbiamo dato la disponibilità ad affrontare la questione con la massima serietà e la dovuta chiarezza, convinti dell'assoluta necessità di percorrere un cammino di normalizzazione del settore. Ma siamo stati altrettanto chiari nel sottolineare che chiudere una vicenda così annosa, complicata e sofferta non poteva rappresentare per noi un obiettivo a prescindere: a prescindere dal rispetto della legge, a prescindere dal riconoscimento effettivo di quegli agricoltori (e sono più del 90 per cento) che hanno obbedito alle regole e che considerano giustamente intollerabile vedersi scavalcare da chi ha sistematicamente eluso le norme. A prescindere, insomma, dai princìpi di legalità, di giustizia, di equità, che devono sempre rappresentare il faro della nostra azione legislativa. Nel corso dell'audizione svolta in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare abbiamo ascoltato i presidenti delle associazioni sindacali di categoria che, con grande serietà e correttezza, hanno illustrato i contenuti dei loro emendamenti. In quell'occasione, venne lanciato in modo evidente un messaggio univoco: rispetto della legalità, trasparenza, chiarezza, equità e su questa base comune erano costruite le diverse proposte emendative. Un atteggiamento propositivo che ha caratterizzato anche i vari incontri tenuti dalle stesse associazioni sui territori ai quali, come parlamentari, siamo stati tutti chiamati. E i medesimi concetti, del resto, hanno contraddistinto anche il documento unitario delle Regioni che, all'unanimità, indipendentemente dal proprio colore politico, hanno espresso il loro parere negativo sui contenuti del decreto, decreto, denunciando come proprio le Regioni siano state espropriate di una prerogativa che la legge sulle quote riserva loro. Altro che federalismo! Per una strana logica del contrappasso questo Governo, anche stavolta come in altre occasioni, si sta dimostrando il Governo più centralista degli ultimi anni. anni. È impressionante il numero di ordini del giorno approvati dai consigli provinciali e comunali che chiedono una revisione del testo del provvedimento; ordini del giorno presentati in molti casi, paradossalmente, da esponenti della vostra stessa maggioranza, che nei nostri territori stanno esprimendo quotidianamente il loro sostegno e la loro solidarietà alla protesta. Ma allora - viene da chiedersi - questo movimento, così incredibilmente trasversale, ha forse preso un abbaglio? Stanno forse tutti dicendo bugie, stanno facendo disinformazione o speculazione politica, come lei ha avuto modo di dichiarare? Nessuno ha letto bene il decreto e gli emendamenti? Sinceramente, signor Ministro, mi sembra per lo meno fuori luogo una lettura così presuntuosa di quanto sta avvenendo nei territori in modo così corale. Ma crede veramente che i nostri agricoltori e i nostri allevatori non siano in grado di leggere bene tra le righe di un provvedimento e capirne le ricadute e le conseguenze? Proprio loro, che in tutti questi anni hanno vissuto sulla loro pelle con fatica, con enormi sacrifici, con investimenti ingenti per stare all'interno delle norme e delle regole. Vengo da una terra - la provincia di Cremona - che ha nel settore della zootecnia da latte uno dei suoi punti di maggior pregio e forza e che, insieme alla provincia di Brescia, è tra i primi produttori di latte dell'intero Paese: il 10 per cento dell'intero quantitativo nazionale viene prodotto nelle nostre province. Ma il prezzo pagato è stato altissimo. In soli dieci anni le aziende zootecniche a Cremona hanno subito una riduzione significativa: da 1.500 insediate nel 1998, il numero aziende che hanno agito nella piena legalità, nel rispetto delle regole, accendendo molto spesso mutui consistenti che pesano sui bilanci aziendali. Come non vedere e non capire che sarebbe inaccettabile e inqualificabile per tutti loro - ma anche per tutti noi far passare il messaggio che si scherzava, che proprio loro rischiano di essere penalizzate e mortificate, mentre la quarantina di aziende sul territorio cremonese, che in modo sistematico hanno splafonato sui grandi numeri, potrebbero avere la meglio? Le assicuro, signor Ministro, che la nostra gente sa benissimo di cosa stiamo parlando, ha letto benissimo cosa c'è scritto nel decreto-legge e ne ha seguito tutte le fasi, da quella iniziale agli emendamenti approvati in Commissione. Sa che il testo del provvedimento è stato modificato in alcune parti, ma che rimane tuttora largamente insufficiente per rispondere a quei princìpi di equità e giustizia di cui parlavo all'inizio; sa che i punti qualificanti del decreto, quei punti che per ora ancora non ci sono (il ritiro dei contenziosi, un'adeguata quantificazione del fondo per gli interventi nel settore, una definizione chiara delle priorità di assegnazione delle quote, la certezza che non siano premiati i furbi), quei punti che tutti stiamo chiedendo con forza - noi, come Gruppo del Partito Democratico con i nostri emendamenti, e gli allevatori nelle loro iniziative - sono punti che fanno la vera differenza, la differenza sostanziale che corre tra la regola e il caos, tra la giustizia e l'iniquità, tra l'onestà e la furbizia. Noi non abbiamo dubbi da che parte stare. Mi auguro perciò che nelle prossime ore, in sede di discussione in quest'Aula, possano essere presi in debita considerazione gli emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato e che sono stati così bene illustrati dal senatore De Castro, volti a colmare quelle lacune ancora per noi presenti, la risposta alle quali determinerà il nostro atteggiamento di voto finale.

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, tante erano e tante sono le aspettative riposte sul decreto che oggi discutiamo in quest'Aula, non solo da parte dei produttori di latte, ma anche da parte dell'intero Paese, e questo non a caso. Infatti, l'attenzione dei cittadini su un provvedimento che appare così fortemente specialistico indica in modo chiaro come il Ministro abbia voluto in modo deliberato concentrare la propria comunicazione su un settore così ristretto per distoglierla dalla mancanza di politiche generali di rilancio dell'agricoltura, che versa oggi in una situazione di gravissima difficoltà. Di ciò il Partito Democratico è consapevole e per questo sta cercando di dettare l'agenda al Governo, presentando una mozione che contiene importanti spunti di discussione e abbracciando analisi e proposte di più lungo respiro rispetto ad un processo di decretazione che ha solo aumentato le incertezze degli operatori del settore. La discussione comunque stimolata ha però fatto emergere la reale portata del provvedimento. Questo, infatti, tocca princìpi e valori più generali, come l'equità, la giustizia, la legalità, che travalicano il tentativo e la fretta di chiudere la vicenda. Questo non è accettabile, non solo per i produttori direttamente interessati che hanno operato secondo le regole, ma anche per il Paese. Non è accettabile una soluzione che si limiti a rendere meno amara la pillola a chi avrà in questa proposta l'ultima inderogabile via di rientro nei meccanismi di distribuzione delle produzioni a cui sono assoggettati i Paesi europei. La definitiva regolamentazione delle produzioni nazionali di latte deve porre fine a tutte quelle distorsioni che l'applicazione delle norme comunitarie in materia ha prodotto in una parte degli allevatori nel corso di questi anni, ponendo il nostro Paese al centro di una procedura a tutt'oggi non conclusa, che ha provocato danni economici e di immagine all'Italia. Quando gli eventi si protraggono a lungo nel tempo si rischia di perdere di vista le cause che li hanno provocati e di costruire soluzioni miopi rispetto al passato, ma che necessariamente lo diventano anche rispetto agli esiti futuri, se queste sono fondate su elementi incerti e non condivisi. I contenuti del decreto evidenziano questa miopia. Esso appare un tentativo di mettere una pietra tombale sul passato, senza tenere conto fino in fondo dei diversi comportamenti tenuti dai produttori,

Purtroppo, l'eccessiva tecnicalità degli articoli rende la lettura dei non addetti ai lavori molto complicata; questo comporta il rischio che, nel tentativo di renderli più semplici, si giunga ad un'interpretazione che viene letta come demagogica, ma che non è tale e che non deve esserlo. Lo sforzo che dobbiamo fare per chi ci ascolta è proprio quello di far emergere in modo chiaro gli elementi principali e pericolosi contenuti nel decreto. Questo è possibile se si parte dalla *ratio* della norma: il ripristino della legalità. Pur nella complessità, risulta chiaro che, tra gli oltre 40.000 produttori, c'è chi ha accettato i meccanismi prodotti dalla normativa comunitaria e nazionale, da subito o aderendo alla legge n. 119 del 2003 che dava a tutti la possibilità di sanare la propria posizione, e chi a tutt'oggi quelle regole non ha mai accettato, avviando e continuando a sostenere contenziosi che sono un chiaro segnale della non disponibilità a rientrare in questo percorso. C'è quindi chi ha sostenuto sacrifici economici, investendo per l'acquisto e per sanare la propria posizione, e chi invece ha continuato a produrre scaricando sugli altri produttori e indirettamente sull'intera collettività i relativi oneri. Se noi non partiamo da questo rischiamo veramente di cadere dalla padella nella brace, vanificando il lavoro fatto e le buone intenzioni delle parti, e io credo che l'unico modo per ridare credibilità al settore ed autorevolezza al legislatore sia quello di definire modi e forme che redistribuiscano diritti e doveri secondo equità. Dalla lettura del decreto il Partito Democratico ritiene che questo si sostanzi in tre modifiche al testo che sono per noi irrinunciabili. La prima è quella di attribuire le quote secondo un ordine che privilegi i comportamenti virtuosi, per cui è sbagliato porre sullo stesso piano coloro che per cercare di produrre in regola sono ricorsi anche all'affitto delle quote e coloro che non hanno mai accettato il sistema, ponendosi in una posizione sleale rispetto agli altri. La seconda è quella di creare le condizioni per cui chi non ha pagato lo faccia, e ciò è possibile solo se l'assegnazione delle nuove quote viene subordinata alla regolarizzazione da parte dell'azienda della propria posizione, rinunciando in via preventiva ai contenziosi avviati, come accadde per chi si regolarizzò nel 2003. luogo, è necessario ripristinare con le risorse versate un fondo da destinare al sostegno degli investimenti effettuati dalle aziende che hanno acquistato le quote, fondo che sia dignitoso e compatibile rispetto agli sforzi fatti dai nostri produttori. Questi sono i punti per noi irrinunciabili; sono richiesti dagli allevatori scesi in piazza, ma anche dal nostro Paese, che, signor Ministro, non riesce proprio a capire perché lo Stato si preoccupi di più delle delle inaccettabili ragioni di quella minoranza che, per anni, ha prodotto in modo irregolare. Le proposte emendative del Partito Democratico accolte in Commissione non sono sufficienti a compensare il rifiuto di modificare questi punti più generali. Mi auguro che la discussione in Aula consenta a lei, signor Ministro, e alla sua maggioranza di rispondere in modo positivo ridando pace al settore e fiducia al Paese. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, lo dico senza mezzi termini: il decreto così come approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 gennaio è uno schiaffo in faccia a tutti quegli agricoltori che in questi ultimi anni hanno prodotto il latte nel rispetto delle norme. Pur di rispettare la normativa sulle quote e restare nella legalità, centinaia e centinaia di produttori hanno contratto mutui e fatto grandi sacrifici. Le recenti manifestazioni contro le nuove norme sulle quote latte - cito testualmente la dichiarazione del presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni, che sottoscrivo pienamente - «sono la risposta civile, pacifica, ma ferma, della legalità che si oppone all'illegalità». Centinaia di produttori hanno dunque giustamente manifestato per ribadire con forza che i furbi non vanno premiati. Oltre a ciò, ci lascia assai perplessi che un Ministro, che per definizione dovrebbe essere federalista, non abbia consultato le Regioni durante l'elaborazione del provvedimento, espropriandole quindi di una prerogativa che la legge sulle quote riserva loro. Signora Presidente, cari colleghi, pur riconoscendo che in Commissione agricoltura sono state introdotte importanti modifiche migliorative che illustrerò tra breve - annuncio fin d'ora che, per i motivi testé ricordati, voteremo contro questo provvedimento per dare un segnale forte e di incoraggiamento a tutti gli agricoltori che in questi anni hanno deciso di stare dalla parte della legge. Come rappresentante del mio Gruppo in Commissione agricoltura, mi permetto ora di illustrare brevemente i miglioramenti dall'esame in Commissione. Innanzitutto, vorrei evidenziare l'importanza di aver inserito nel testo un esplicito riferimento alle zone montane, con ciò includendole fra le realtà svantaggiate ed evitando una disparità di trattamento. Tengo a sottolinearlo perché reputo assai importante dare un segnale di sostegno a queste aree, viste le enormi difficoltà che gli agricoltori di queste zone si trovano a dover fronteggiare. È noto che le zone montane soffrono di svantaggi che rendono questa agricoltura meno facilmente adattabile alle condizioni di concorrenza Oltre ai problemi geomorfologici, l'agricoltura delle zone montane deve affrontare soprattutto svantaggi climatici che influenzano la normale tecnica agronomica e zootecnica delle aziende e incidono in misura significativa sui costi e sulle strategie aziendali. Questo è anche uno dei motivi esplicativi del fatto che queste zone sono caratterizzate da scarsa densità e oggi, purtroppo, persino dalla tendenza ad una regressione demografica.

Ringrazio poi la Commissione per aver accolto una nostra richiesta a sostegno delle assicurazioni antigrandine. Fino al 2008, infatti,

con 330 milioni per l'anno 2009 e con 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Infine, ringrazio per aver accolto una richiesta avanzata ossia la proroga fino al 31 dicembre 2009 della disposizione sulle agevolazioni previdenziali previste dalla legge n. 205 del 2008, in favore degli imprenditori agricoli ubicati nelle zone montane particolarmente svantaggiate.

Non è questa la sede per una puntuale ricostruzione storica della vicenda delle quote latte. Tuttavia, poiché, quella appena fatta è una affermazione decisamente forte, riteniamo necessario ricordare alcuni momenti particolarmente significativi che, nel loro insieme, dimostrano come in questo Paese, dal 1984 al 2003, l'obbligo del rispetto del regime comunitario delle quote latte sia stato, di fatto, disatteso. Ci vogliamo, in particolare, riferire, ai fatti seguenti: subito dopo la prima applicazione, nel 1987, quando vigeva la figura del produttore unico che, in Italia, era rappresentata dalle Unioni, l'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnò a tali soggetti una quota complessiva superiore del 5 per cento rispetto a quella che la CEE aveva attribuito al nostro Paese. Nel 1991, una legge dello Stato, la n. 201 del 10 luglio, all'articolo 1, comma 3, disponeva: «Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca si applicano a partire dal periodo 1991-1992 su tutto il territorio nazionale», riuscendo così, in un colpo solo, a derogare ad un obbligo sancito dalla Costituzione (il rispetto dei regolamenti comunitari) e a cancellare, di fatto, sette anni di partecipazione dell'Italia alla CEE, in quanto, come noto, le quote latte erano in vigore dal 1984 e non dal 1991-1992. 1991-1992. La legge n. 468 del 26 novembre 1992, che pure avrebbe dovuto garantire il rispetto delle regole comunitarie, assegnava ai produttori non una quota, ma due: la quota la quota A, che corrispondeva a quanto prodotto e commercializzato nel 1988-89, e la quota B, che rappresentava l'incremento produttivo rispetto alla quota A, che era stato irregolarmente realizzato fino al 1991-92 e che, pertanto, avrebbe dovuto essere linearmente ridotto a tutti i produttori, al fine di rientrare nei limiti della quota assegnata dalla Comunità. Quota B che, invece, come ben sappiamo, fu ridotta non a tutti, ma solo ad alcuni, creando un problema, con le cui stratificazioni siamo, ancora oggi, costretti a fare i conti, ogni qualvolta si legifera in materia di quote latte. Nella XIII legislatura, i quattro Governi di centrosinistra che si alternarono alla guida del Paese emanarono ben undici decreti-legge in cinque anni, per apportare ripetute modifiche alla legge n. 468 del 1992, complicandone i già discutibili contenuti, al punto da renderli, di fatto, inapplicabili; come, inequivocabilmente, dimostravano gli oltre 20.000 ricorsi aperti contro AGEA che, alla fine della stessa legislatura, risultavano essere stati avanzati da parte dei produttori. In questo quadro a dir poco devastante, nella XIV legislatura, il Governo di centrodestra riuscì, per la prima volta dal 1984, a mettere a punto un nuovo quadro normativo nazionale che garantisse l'applicazione del regime delle quote latte in condizioni di legittimità e di certezza del diritto. Ciò è accaduto con la legge n. 119 del 2003 che, non a caso e contrariamente a quanto accaduto per le norme nazionali del passato, è rimasta invariata fino ad oggi. Questa breve ricostruzione si è resa necessaria proprio per dare rilevanza al fatto che, nel 2003, per la prima volta dopo venti anni, l'Italia si è dotata di una norma nazionale che ha consentito - e continua a consentire - la corretta applicazione del regime delle quote latte. Una norma che era e resta valida anche oggi a seguito dell'emanazione del decreto-legge che siamo chiamati a convertire. È questa una precisazione importante che consente di sgomberare il campo da alcune delle tante strumentalizzazioni che, da più parti, si stanno facendo e che, nel caso specifico, cercano di far passare il presente decreto-legge come un provvedimento che mette in discussione l'impianto della legge n. 119 del 2003, delegittimando l'intero quadro normativo nazionale, in materia di quote latte. Si tratta, come dicevamo, di vere e proprie strumentalizzazioni, finalizzate a confondere le idee riguardo all'effettiva natura del presente decreto-legge che - giova ribadirlo con chiarezza non è un provvedimento che altera le regole, ma è un provvedimento che interviene per assicurare l'equa e corretta gestione di un fatto straordinario e straordinariamente positivo, rappresentato dall'assegnazione delle quote ottenute dal ministro Zaia, nell'ambito del recente negoziato comunitario del cosiddetto Dal 1984 in avanti, il problema della mancata applicazione delle quote latte ha inciso negativamente sulla credibilità dell'Italia nelle sedi comunitarie. Il fatto stesso che, dopo innumerevoli tentativi, la Commissione UE sia arrivata alla determinazione di concederci un significativo aumento di quota è, in primo luogo, una grande apertura nei confronti dell'attuale Governo, cui va il merito di essere stato ritenuto credibile proprio sul terreno in cui la credibilità dell'Italia era, storicamente, tendente a zero. L'aumento di quota è stato un grande successo, i cui meriti sono indubbiamente da riconoscere al ministro Zaia. Tale successo non è però un alloro sul quale riposare felici e spensierati ma costituisce, come ho detto, un riconoscimento di credibilità e, proprio per questo, si fonda sull'obbligo di confermarci credibili. Come ben sappiamo, l'aumento di quota non ci è stato concesso a fondo perduto per poter accrescere la nostra produzione di latte senza rendere conto a nessuno. Su questo punto occorre essere ben chiari. Le nuove quote non possono e non devono essere impiegate per produrre di più, ma sono unicamente da destinare al riassorbimento degli attuali surplus produttivi per impedire che si formino nuove multe nei sei anni che ci separano dalla scadenza del regime delle quote latte e affinché a tale scadenza le nostre imprese possano arrivare in condizioni migliori di quelle in cui ci troviamo adesso. È evidente che,

In questo senso, i problemi da affrontare erano molti e complicati. Vi era da garantire l'equità della distribuzione delle nuove quote e da evitare che si creassero situazioni di svantaggio per coloro che avevano sempre rispettato le regole o di favore per chi non è stato altrettanto virtuoso o, addirittura, si è posto volontariamente al di fuori del sistema. Vi era anche da cogliere l'opportunità veramente straordinaria dell'aumento delle quote che, per la prima volta, consentiva non solo di uscire dal tunnel delle multe certe alla fine di ogni campagna, ma anche di ricondurre nell'alveo della regolarità tutte le imprese che per vari motivi ne erano uscite. Per risolvere questi difficili problemi era necessario un provvedimento rigoroso, quale certamente è il decreto-legge che siamo chiamati a convertire. Tuttavia, come ben sappiamo, le risposte rigorose ai problemi difficili, proprio perché destinate ad essere risolutive, non sono gradite a coloro che, dall'esistenza e dal perdurare dei problemi storicamente irrisolvibili, hanno tratto e traggono linfa vitale per alimentare la loro presenza e, in alcuni casi, la loro rappresentanza. Ed è probabilmente proprio per difendere interessi corporativi, che sono destinati a venire meno a seguito della risoluzione dei problemi di cui fino ad oggi si sono alimentati, che, da più parti, si stanno verificando così tante strumentalizzazioni contro il presente decreto-legge. In particolare, si sente dire che con questo provvedimento non si rispettano coloro che hanno sempre osservato le regole e che si assegnano quote ai cosiddetti splafonatori di professione; che si attua una vera e propria sanatoria in favore di coloro che si sono rifiutati di riconoscere e, quindi, di pagare gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare; che si fa perdere valore alle quote acquistate nel recente passato e si creano le condizioni per nuove riduzioni del prezzo del latte e, quindi, per un'ulteriore perdita di competitività del settore. Sembra quasi impossibile che tali strumentalizzazioni possano avere luogo a fronte di un testo i cui contenuti sono molto chiari e facilmente leggibili. Eppure, questa è la realtà

Eppure, questa è la realtà con cui oggi siamo chiamati a confrontarci. Per tale motivo, anche al fine di recare un contributo al sereno esame del provvedimento da parte di quest'Aula, in primo luogo, che non vi è alcuna discriminazione in favore dei cosiddetti splafonatori di professione, tanto è vero che le quote saranno assegnate solo agli allevatori in produzione ed unicamente per coprire i surplus produttivi realizzati nel 2007-2008, al netto delle quote vendute dal biennio 1995-1996 in avanti. segno evidente che obiettivo chiarissimo e - oseremmo dire - chirurgico del presente decreto è quello di evitare che si producano quantità aggiuntive di latte e, quindi, di andare a destinare le nuove quote unicamente a riassorbire i quantitativi che hanno dato origine a multe, affinché le stesse non compaiano più fino alla scadenza, nel 2015, del regime comunitario delle quote. Allo stesso modo non è assolutamente vero che saranno solo i 4.260 splafonatori a beneficiare delle nuove assegnazioni che, invece, sulla base delle priorità indicate nel decreto, si distribuiranno tra ben 17.000 imprese, ossia interesseranno il 42,5 per cento delle aziende in produzione. In secondo luogo, ribadiamo che non vi è alcuna sanatoria per le multe pregresse, la cui restituzione avviene dietro pagamento di rate gravate di un tasso di interesse che di fatto è pari a quello che, a parità di durata, chiunque può spuntare in una banca per un mutuo a tasso fisso. Si tratta pertanto di una restituzione di un debito ad un tasso che non è esagerato definire di mercato. Le sanatorie, come è noto, sono ben altro. Anche questo aspetto costituisce un'ulteriore prova che non vi è alcuna discriminazione nei confronti di coloro che nel 2003 decisero di mettersi in regola e che beneficiarono di una rateizzazione che, essendo senza interessi, era indiscutibilmente assai più favorevole di quella contenuta nel presente decreto. Ma non solo, l'accettazione e, quindi, il pagamento degli importi pregressi imputati a titolo di prelievo supplementare è la condizione indispensabile per avere accesso all'assegnazione delle nuove quote. I contenuti del decreto, al riguardo, sono tanto chiari quanto intransigenti: solo chi si mette in regola e rispetta le scadenze dei pagamenti può accedere alle nuove assegnazioni e conservarle. Come si vede, è una realtà ben diversa da quella che da più parti si vorrebbe far apparire. Così come totalmente infondate e strumentali sono quelle teorie che cercano di mettere in relazione le nuove assegnazioni con la perdita di valore delle quote la riduzione dei prezzi che dovrebbe verificarsi a seguito di un ipotetico aumento della produzione, a sua volta conseguente all'attribuzione dei nuovi quantitativi. La perdita di valore delle quote è un fatto inevitabile, che non è conseguente alle nuove assegnazioni, ma al fatto che è ormai certa la scadenza del regime delle quote latte. È infatti evidente che, con l'approssimarsi della data del 31 marzo 2015, le quote vedranno, progressivamente, ridursi il loro valore, finché lo stesso evaporerà del tutto. È questo un processo inevitabile e del tutto fisiologico, sul quale le nuove assegnazioni non avranno, né potranno avere incidenza alcuna. Altrettanto pretestuosa ed infondata è la teoria che le nuove assegnazioni determineranno un aumento di produzione che, a sua volta, provocherà un'ulteriore riduzione dei prezzi, aggravando la già pesante situazione in cui versa il comparto. La flessione dei prezzi è in atto da tempo e ha le sue ragioni non nelle quote che, anzi, avendo assicurato un diritto a produrre, il prezzo l'hanno difeso, ma in cause strutturali, che vedono la componente agricola e di trasformazione perdere peso e potere contrattuale nei confronti della distribuzione, alla quale ormai va circa il 60 per cento del valore che si produce, a fronte del 23 per cento e del 17 per cento che vanno, rispettivamente, all'industria e all'agricoltura. Non si capisce, pertanto, come il presente decreto possa negativamente incidere su dinamiche da tempo in corso, nonché dipendenti da tutt'altre cause. Tanto più che i contenuti del decreto sono rigorosamente finalizzati ad utilizzare le nuove assegnazioni per riassorbire le attuali eccedenze e, quindi, ad evitare che le stesse si ad evitare che le stesse si trasformino in produzioni aggiuntive ed in ulteriori multe. D'altronde, non si capisce per quale motivo il Governo dovrebbe perseguire un obiettivo diverso, non solo da quello che dichiara, ma anche da quello a cui è tenuto per il rispetto delle condizioni in base alle quali la Commissione europea ci ha concesso le quote aggiuntive e che - giova ricordarlo - prevedono che il superamento dei nuovi quantitativi comporti il pagamento di un prelievo maggiorato del 150 Anche questo è un modo attraverso il quale, da un lato, la Commissione europea ha inteso misurare la nostra credibilità e, dall'altro lato, il nostro Governo intende dimostrare di essere credibile. Anche per questo siamo convinti che, come già detto, il presente decreto costituisca una risposta rigorosa ad una serie di problemi difficili e che, pertanto, meriti di essere convintamente sostenuto, non solo per assicurare il futuro sviluppo del nostro settore lattiero-caseario, ma anche per l'immagine dell'Italia, che riesce a mettere definitivamente ordine in una questione che, per 25 anni, è stata sistematicamente e strumentalmente utilizzata nelle sedi comunitarie come l'emblema della nostra scarsa credibilità.

*(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi presenti in quest'Aula, stiamo discutendo di un provvedimento che, è bene chiarire subito (lo hanno fatto i senatori che mi hanno preceduto), va definito per quello che è, ovvero un condono a favore delle poche, anzi pochissime aziende - e lo sottolineo - che, in spregio alle regole dell'Unione europea e al dettato normativo della legge n. 119 del 2003, si sono mosse nella illegalità, e non garantisce minimamente i tanti,

Mi chiedo come si possa negare l'evidenza in merito, quando, secondo diversi calcoli, gli splafonatori che hanno generato il 75 per cento dei 168 milioni di euro per il superamento delle quote latte sarebbero appena 646, a fronte di 41.000 produttori: sono dati pubblicati dalle organizzazioni, caro signor Ministro. E anche qui, rispondendo al collega che mi ha preceduto, voglio ripetere che il negoziato che ha assegnato all'Italia un ampliamento delle quote del 5 per cento, ha concesso di farlo in maniera anticipata con un preciso obiettivo: stabilizzare il mercato, sanando le irregolarità. Di questo stiamo parlando. Ciò premesso, vorrei rassegnare alcune considerazioni su questo decreto. In primo luogo, sarebbe stato preferibile applicare una legge già vigente, perché la legge c'è (lo dico sempre e voglio parlava prima di confusione legislativa: quindi, non è colpa loro, se non hanno pagato, mentre tutti gli altri l'hanno fatto, caro collega): mi riferisco alla legge n. 119 del 2003, votata all'epoca da gran parte della maggioranza e dell'opposizione, dal momento che in tempi anche recenti ha prodotto buoni esiti. Inoltre, mi sembra opportuno sottolineare che, contrariamente a quella buona legge che individuava nelle Regioni gli organi deputati all'amministrazione delle quote dei rispettivi territori, questo decreto non le coinvolge minimamente nella modalità di ripartizione delle quote nel territorio nazionale; e questo, se permettete, cari colleghi, appare quantomeno singolare, da parte di un Governo, di un Ministro e di una forza politica che spingono sul federalismo, e dunque sul protagonismo delle Regioni e dei poteri locali, con un decisionismo centralista senza precedenti. Vorrei sottolineare, signora Presidente, signor Ministro, che il Partito Democratico ha seguito tutto l'*iter* del provvedimento in Commissione agricoltura, con un atteggiamento, tra l'altro, costruttivo e collaborativo, ma tutte le proposte di modifica, ampiamente condivise da larga parte del mondo produttivo, sono state respinte. Il provvedimento, come sappiamo e come abbiamo dichiarato in questi giorni, è largamente al di sotto delle aspettative del Partito Democratico e degli stessi operatori che stanno manifestando in piazza, con una forte e civile

paghi tutti gli arretrati e rinunci ai contenziosi giudiziari, almeno la prima rata del 2009. Questo è un punto irrinunciabile che il Partito Democratico

perché si riferisce a debiti esigibili e chiunque di noi abbia fatto semplicemente l'amministratore locale sa che questa norma non si può certo applicare ai contenziosi in Io qui, signor Ministro, non vorrei pensare male, ma dal 2014, come ha detto stamattina in un'intervista, le quote saranno abolite: basterà rinviare con qualche furbizia i pagamenti ed ecco che le multe non si pagheranno. Credo che questo non sia affatto giusto. sia affatto giusto. L'altro punto per noi irrinunciabile era invertire l'ordine di priorità di assegnazione delle quote. Lo stesso Fondo che avete aumentato di 10 milioni di euro non servirà a risolvere il problema né a stemperare la tensione e le preoccupazioni degli allevatori.

Ha contestato questo principio, dicendo che sono stati tagliati i fondi a tutti i settori e invece io le ho ricordato molto semplicemente

lo stesso Ministro di questo settore ritenga che il comparto primario, che ovviamente ha una parte consistente nella bilancia *import-export* e nel nostro prodotto interno lordo, abbia una priorità in questo Governo. Per noi del Partito Democratico l'agricoltura e l'agroalimentare hanno precise priorità in questo Paese e in un momento di crisi di questo Paese, caro Ministro.

Noi ancora una volta siamo disponibili affinché il decreto al nostro esame venga modificato, ma lo facciamo soprattutto se da parte di questo Ministro e della Commissione vi è un atteggiamento di serietà e soprattutto di grande apertura, che non mi pare abbia mostrato in questi giorni.

noi siamo dalla parte dei tanti allevatori onesti e siamo per una battaglia per la legalità, per il rispetto delle regole, principi imprescindibili per una libera concorrenza e una sana competitività in questo Paese.

Signora Presidente, signor Ministro dell'agricoltura, onorevole Zaia, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è volto a disciplinare rilevanti profili in tema di quote latte

sono oggetto da anni di svariati tentativi allo scopo di individuare un punto di equilibrio tra gli interessi dei produttori e i limiti stabiliti dall'Unione europea, che hanno comportato l'applicazione di sanzioni di una grande entità. Il negoziato condotto dal Governo Berlusconi nella persona del ministro Zaia, in sede europea, consente peraltro di riconsiderare in una chiave migliore tutti gli aspetti della vicenda, dal momento che l'Italia ha ottenuto,

Dalla ripartizione di tali quantitativi, che ammontano a 757.000 tonnellate, deriverà una situazione di equilibrio tra quote e produzione, in modo da evitare gli esuberi che hanno caratterizzato l'applicazione del regime delle quote nel nostro Paese. Per questo aspetto, il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura, egregiamente condotto dal presidente, senatore Scarpa Bonazza Buora, ha introdotto importanti modifiche in base alle quali, mantenendo la priorità a favore delle aziende con quota B ridotta ed effettivamente prodotta, si prevede l'assegnazione delle nuove quote anche alle aziende ubicate in zone montane, e, soprattutto, coloro che hanno coperto gli esuberi produttivi mediante gli affitti vengono collocati sullo stesso piano dei produttori eccedentari. Con tali scelte saranno ricomprese nella ripartizione una parte rilevante delle aziende attualmente in attività, pari a circa 17.000 su un totale di circa 40.000 allevatori, coprendo perciò il 42,5 Si fa presente, peraltro, che sono più di 8.000 le aziende che dovranno pagare per un totale di circa 1 miliardo e 670 milioni di euro e tra queste circa 4.200 aziende sono ancora in attività e producono circa il 25 per cento del latte italiano. Inoltre, la Commissione agricoltura ha previsto che il Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, con la dotazione di 25 milioni di euro con il ricorso a precedenti stanziamenti agricoli, sia destinato prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte, sviluppando, per un effetto moltiplicatore, un importo di 250 milioni di euro, da utilizzare, mediante il rilascio di garanzie pubbliche a prima richiesta, per la ristrutturazione dei debiti derivanti dalle operazioni di acquisto o per facilitare l'accesso al credito. In relazione al recupero delle multe pregresse è stata prevista una procedura di rateizzazione onerosa, pur se diluita nel tempo; i soggetti ammessi alla procedura dovranno pagare rate con interessi

Gli emendamenti approvati dalla Commissione agricoltura sono stati finalizzati a porre maggiori vincoli e regole più precise, rispetto al testo originario del decreto-legge, in modo da assicurare l'adempimento degli obblighi assunti. Al riguardo, chi non si metterà in regola avrà il blocco degli aiuti fino a quando non avrà saldato il suo debito e se sarà insolvente perderà le quote assegnate ed in caso di sovrapproduzione la sanzione aumenterà del 150 A differenza di valutazioni frettolose, spesso dettate da un approccio pregiudiziale o da disinformazione, si ritiene che il provvedimento vada incontro alle attese degli allevatori

altre questioni fondamentali che affannano tutto il settore agricolo. Tra queste ricordo solo per un momento la inefficienza della filiera e l'enorme divario fra il prezzo alla stalla e quello al consumo. Più in generale, si è in attesa di provvedimenti che prorogano le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate e contemplano il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la copertura dei premi assicurativi avverso le calamità naturali; emendamenti che, peraltro, sono stati approvati in Commissione agricoltura e che attendono oggi il vaglio della Commissione bilancio. *(Applausi

un atto amministrativo - non voglio qui illustrarlo - che creava delicati problemi di restituzione di 11 milioni di euro a 915 famiglie per un contenzioso amministrativo; dell'assegnazione di 14 milioni di euro decisi dal Ministero della difesa, che però non sono arrivati al corpo militare della Croce rossa italiana; infine, il problema di 378 militari richiamati, precari da un decennio, che sono stati esclusi dalle procedure di stabilizzazione previste dalle recenti leggi finanziarie. Poiché in Commissione difesa stiamo discutendo di disegni di legge quale quello relativo all'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al corpo militare della Croce rossa italiana (quindi con un potenziamento ed una valorizzazione del ruolo),

Grazie